Dobbiamo ricordare ciò che ieri ha riferito il Ministro: il processo civile telematico è attivo con valore legale per i decreti ingiuntivi in 25 tribunali, in 12 per l'esecuzione, in 8 per il settore fallimentare e in 5 per i pagamenti elettronici. Basti pensare che a dicembre 2008, a fronte di un investimento di 600.000 euro, non vi era alcuna di queste attività svolte in nessuno dei tribunali italiani.

attivo il sistema *web* di gestione dei registri informatici per la cognizione ordinaria, così intendo ricordare che la consultazione via Internet dei dati e documenti personali è stata realizzata in 157 tribunali su 165. Mi limito soltanto a citare alcuni degli esempi riportati nella relazione del Ministro, come ad esempio la consultazione evoluta da parte degli avvocati che è attiva in 10 corti di appello e 89 tribunali. per dimostrare che in questi due anni vi è stata un'accelerazione nel sistema di informatizzazione che ha portato a quella diminuzione che il Ministro ieri ha citato come primo dato e il senatore D'Ambrosio correttamente ha evidenziato che bisogna tener conto anche di quali sono le sopravvenienze. a una diminuzione della pendenza di 223.824 procedimenti e che tiene conto di un ulteriore dato: negli ultimi 10 anni l'aumento della pendenza era di 200.000 procedimenti annui. Quindi non solo non c'è stato per la prima volta l'aumento di 200.000 procedimenti, ma la diminuzione di oltre 223.000. sono la riforma del processo civile, l'informatizzazione degli uffici giudiziari, la modifica in tema di spesa di giustizia e in particolare - questa è parte della relazione la disciplina del contributo unificato, che ha ridotto sensibilmente il numero delle opposizioni alle sanzioni amministrative, determinando una diminuzione delle sopravvenienze e una capacità di solerte e proficuo lavoro dei magistrati. Questa è stata l'indicazione del Ministro sulla base dei dati raccolti. Nel penale vi è stata una diminuzione della pendenza di circa 45.000 procedimenti.

dei filoni d'intervento che possano trovare consenzienti e d'accordo maggioranza e opposizione. Poi ci si può dividere su singoli provvedimenti, su singoli aspetti, ma sulla questione generale credo che ciascuno di noi dovrebbe fare uno sforzo.

a riformulare l'emendamento del senatore Vizzini tenendo conto di utili indicazioni che venivano dagli emendamenti dei senatori Lumia e D'Alia, D'Alia, rinunciammo come Governo a presentare la riformulazione dell'emendamento sul 41-*bis*, che, fatto proprio dal senatore Vizzini, fu sottoscritto dai senatori Lumia e D'Alia determinando un'approvazione all'unanimità. Pertanto il Governo, nonostante avesse contribuito all'elaborazione del provvedimento, ha rinunciato a presentarlo. Ritengo che questa dovrebbe essere la tecnica, il modo, il comportamento del Governo, dei singoli parlamentari, delle forze politiche per raggiungere dei risultati che sono nell'interesse generale. Poi ci si può dividere su singole soluzioni; si possono interpretare diversamente gli interventi necessari. Però quando abbiamo un progetto, e viene indicata dal Ministro la realizzazione del progetto del *best practice* finanziato dal Fondo sociale europeo per 23 milioni di euro attraverso le Regioni con una programmazione per il 2007-2013 che riguarda 96 uffici giudiziari, queste sono cose che non possiamo negare, ma che tutti dovremmo cercare di valorizzare per individuare

si afferma che non si approva la relazione del Ministro. Lo capisco anch'io, se il dato di fatto a cui ci si riferisce non tiene conto della realtà e si parla ancora della mancanza di fondi per la digitalizzazione e della necessaria copertura per gli ultimi sei mesi; non si tiene conto del fatto, però, che ieri il ministro Alfano ha dato atto di aver risolto il problema per l'intero 2011.

nella relazione del Ministro si indicano procedimenti amministrativi e previsioni non illusorie,

i fondi reperiti, le indicazioni specifiche per le carceri e gli istituti che saranno realizzati, individuando

che nei due anni trascorsi sono stati realizzati 2.250 posti detenuti rispetto alla realizzazione di 2.000 posti detenuti nei dieci anni precedenti: quindi, quello che è stato fatto in dieci anni è stato realizzato in due.

di una pena che serve a redimere il condannato, a ridargli una speranza futura e a reinserirlo nella società si deve in gran parte al sacrificio e alle modalità di gestione della Polizia penitenziaria, in una difficile situazione di sovraffollamento a tutti nota.

il provvedimento di riduzione a tre dei riti civili fondamentali. Ricordo - basta verificare le statistiche, che leggeremo tra qualche giorno anche nelle relazioni dei presidenti di corte d'appello

l'ipotesi di mettere allo studio un provvedimento di amnistia. Nella passata legislatura, quando fu approvato un indulto senza l'amnistia,

particolare, sul primo punto del dispositivo relativo all'informatizzazione e alla distribuzione uniforme dei fondi, revisione delle circoscrizioni, notifiche di atti, di carceri e polizia penitenziaria, mi riporto con riferimento alla Polizia penitenziaria e alle carceri a quanto già detto. Sulla ripartizione dei fondi del Fondo unico giustizia rispetto ai quali si dice che sarebbe opportuno prevedere una maggiore somma da destinare all'amministrazione della giustizia, rilevo che mentre nella norma

che l'intervento sulla mediazione civile è un fatto positivo, si danno indicazioni volte a tener conto delle preoccupazioni degli avvocati, che vorrebbero rinviare.

Quando si parla dei meriti delle forze di polizia e della magistratura specializzata in materia di contrasto alle organizzazioni mafiose, non posso non essere d'accordo, però sarebbe ingeneroso

di dover realizzare norme in materia di lotta alla mafia, norme che hanno portato non solo ad inasprire il 41-*bis* e a prevederne specificamente le condizioni, ma anche quella normativa in materia di sequestri dei beni dei mafiosi che si rivolge anche nei confronti degli eredi, determinando una delle conseguenze più positive nella lotta alla mafia. Non abbiamo mai proposto una limitazione dell'indipendenza del pubblico ministero o la sua sottoposizione all'Esecutivo.

in particolare alla responsabilità del magistrato e al controllo del lavoro da esso svolto. Possiamo essere d'accordo sulla necessità di apportare possibili miglioramenti alla riforma della professione forense e il Governo si impegna ad un costruttivo confronto con tutti i Gruppi parlamentari, sia di maggioranza che di opposizione.

della legge sulle intercettazioni e si tiene conto di emendamenti approvati. Il Governo non può non essere d'accordo

a prescindere che non si tratta di un provvedimento di immediata discussione. Non l'accetto perché il sistema poteva essere corretto. Un fatto è sostenere che una determinata norma può essere corretta per raggiungere determinati risultati; altro fatto è sostenere che, con quella norma, si mandavano al macero determinati procedimenti. In quella occasione, in quest'Aula del Senato, avevo sostenuto che, se di quei processi penali che venivano ad essere eliminati, alla fine del triennio

ringrazio, signor Presidente. del 2005, è sembrata una comunicazione, anche soprattutto in rapporto alla sintesi consuntiva del 2010 fatta dal Ministro e gli orientamenti e i programmi per il 2011. Ne è emerso un chiaro scompenso tra quello che c'è stato nell'anno appena trascorso, quello che, sempre nell'anno appena trascorso, non è stato fatto, e le previsioni su quello che nel 2011 dovremo aspettarci. Abbiamo difatti 28 pagine per il primo punto e poco più di un paio per ciò che ancora c'è da fare. Come dire che sulla giustizia s'è fatto quasi tutto, forse anche che la giustizia funziona bene, e che ci rimane ancora poco per ottimizzarne il funzionamento. Salvo poi, a pagina 29, se non contraddirsi, quanto meno andare in controtendenza rispetto all'impianto di tutta la relazione, riconoscendo il Ministro che una radicale riforma in tema di giustizia non ha visto neppure l'alba e aggiungendo - incredibile - che la colpa di tutto ciò è sostanzialmente da imputare - cito testualmente «all'evoluzione del quadro politico nel secondo semestre nell'anno appena trascorso; le tensioni dell'ultima parte del 2010 hanno ritardato la presentazione in Parlamento di una serie di proposte di legge che continuano a perseguire gli obbiettivi dell'efficienza del sistema giudiziario...». In altri - mi rivolgo al Ministro, che non è presente - imputando proprio a Futuro e Libertà (o - diciamo noi - a chi ne ha causato la sua nascita), imputando al presidente Fini (o - diciamo noi - a chi lo ha cacciato per incompatibilità con i valori del PdL), che la traccia riformatrice della giustizia italiana, forse un po' strabica, continua a mantenere un'attenzione più per il Presidente del Consiglio che per l'interesse generale e preminente di tutti i cittadini. Proprio ieri sera è stato ricordato al Ministro stesso in una trasmissione televisiva come persino nell'ultimo disegno di legge

è, invece, proprio per tutte queste contraddizioni, che la riforma della giustizia, come tutte le altre riforme previste dal programma di Governo, non ha visto se non enunciazioni di principio nei due voti di fiducia che abbiamo avuto a poca distanza tra loro? Le riforme non si fanno perché è sempre colpa degli altri? Stiamo, anzi ora state governando, da 8 anni su 10, e chi oggi come noi non è più in questa maggioranza ha affermato e continua ad affermare

come previsto nel programma elettorale, che ci ha visto eletti insieme (quindi anche una riforma sulla giustizia), siamo disposti a sostenerlo e a votarlo. Basta che, oltre alle relazioni, o alle comunicazioni, come le definiamo noi, queste riforme arrivino in Aula. Devo perciò ravvisare che la relazione del Ministro non è sicuramente improntata, come in altre occasioni invece era avvenuto anche per merito suo, ad una disponibilità al dialogo, all'apertura politica, all'allargamento e alla condivisione dei percorsi politici, riconoscendo, magari, errori di percorso del Governo nella ricerca di un effettivo ampliamento nel nel metodo e nella sostanza di ciò che questo Parlamento, assieme al Governo, può fare per dare risposte concrete al Paese. È un vero peccato, perché è l'ennesima occasione persa per ricucire degli strappi e, dietro a questo atteggiamento di autosufficienza, di autoreferenzialità che tocca, nella relazione di maggioranza del PdL, persino dei toni enfatici, intravediamo senza troppa fatica la solita volontà di alzare una cinta protettiva attorno ai perduranti e oramai asfissianti problemi personali del Presidente del Consiglio rispetto al tema giustizia. Anche sui fatti che in questi giorni vedono coinvolto il Premier, noi ieri mattina abbiamo evitato accuratamente di partecipare all'improvvisato dibattito sull'argomento, dibattito peraltro non previsto dalla che poche ore prima aveva stabilito il calendario, a dimostrazione di non voler cavalcare in chiave politica una vicenda che può solo risolversi e chiarirsi in sede giudiziaria, quando e se - lo speriamo ancora - il presidente Berlusconi deciderà di recarsi dal magistrato, portandoci così a capire se è lui che ha torto o se hanno torto i magistrati che lo hanno inquisito. E mi sembra che a quel dibattito noi di Futuro e Libertà abbiamo seguito la stessa linea del Gruppo della Lega Nord, poco incline in queste ore a rilasciare, come noi, dichiarazioni sull'argomento. Affermare che la riforma della giustizia è stata ostacolata da tensioni politiche che noi avremmo causato, come - ripeto - segna con chiarezza la relazione del Ministro, ci sembra quindi un alibi non degno dello stesso ministro Alfano, che tutti noi stimiamo da sempre. Per smentire quest'affermazione basterebbe misurare il tempo che il Parlamento ha dovuto dedicare a leggi che non miravano affatto ad una riforma del sistema ma a fronteggiare situazioni circoscritte che non interessavano la collettività. È ciò che ci ha ricordato ieri anche la presidente Giulia Bongiorno. Prendendo atto del dato relativo alla riduzione delle pendenze civili, per esempio, anche se, posto che con sempre maggior frequenza esso dipende in realtà dall'abbandono delle azioni stesse, sarebbe utile per il lavoro che qui stiamo facendo verificarne la genesi: non si può infatti escludere che tale abbandono derivi da una crescente sfiducia del cittadino nei confronti della giustizia. A questo proposito, sempre la presidente Bongiorno ieri ci ha anche ricordato come siano significativi i dati diffusi dalla Banca Mondiale nel rapporto *Doing Business* 2011, nella parte dedicata alla giustizia civile e alle procedure per dare attuazione ai contratti. Secondo gli indicatori della Banca Mondiale, che tengono conto anche della lunghezza dei processi civili e dei relativi costi, l'Italia figura al 157° posto su 183 Paesi. Vi è poi il tema delle risorse che ha visto il Ministro in estrema difficoltà, così come, nelle ultime settimane in particolare, nell'identica situazione si sono trovati il Ministro della cultura, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, in quella mannaia metodologica che noi da oltre un anno contestiamo, quando ancora non eravamo costituiti in Gruppo autonomo, cioè quella dei cosiddetti tagli lineari del ministro Tremonti. Sul piano generale noi insistiamo da almeno due manovre finanziarie ad individuare in ulteriori tagli - con un recupero quindi di risorse ulteriori da fare nelle ancora ampie sacche di sperpero nella pubblica amministrazione e nel recupero dei cosiddetti fondi perduti la strategia per andare oltre il contenimento della spesa pubblica, passando così, con il recupero di risorse, alla fase dello sviluppo e del rilancio economico. Ma ricordiamo al Ministro che oggi non c'è, ma ci rivolgiamo al Sottosegretario - che la giustizia, prima che fonte di costi per otto miliardi l'anno, produce molti e forse più euro con confische, prevenzione e repressione dei reati, nonché con la risoluzione delle controversie civili. È giusto quindi che anche da quel Fondo unico giustizia, come chiediamo nella proposta di risoluzione presentata assieme agli amici del Polo della Nazione, si calcolino e si individuino ulteriori risorse per questo settore. risoluzione puntualmente elenchiamo gli ambiti principali di intervento per una riforma seria, non dimenticando soprattutto lo stato emergenziale delle carceri italiane. Al ministro Alfano chiediamo se non siano questi i veri motivi per cui le riforme, anche questa sua sulla giustizia, non si riescono a fare con l'attuale Governo, non certo per le turbolenze politiche che secondo il Ministro avremmo causato noi di Futuro e Libertà in questi mesi. Per trovare i fondi per poter così tamponare l'anno in corso nell'ambito dell'informatizzazione dei tribunali, la sua fatica - glielo riconosciamo - è stata tanta. Ma come possiamo immaginare una programmazione pluriennale in questo settore che non dà né respiro né speranza per l'annunciata riforma? Riforma che noi non ravvisiamo più in questa relazione/comunicazione essere ancora centrale nei programmi di governo. In conclusione, signor Sottosegretario, il nostro voto sarà contrario, prima ancora che per i tanti punti che non ci convincono di questa relazione - nonostante lo sforzo di questa mattina relativamente alla nostra proposta di risoluzione - soprattutto perché con chiarezza voi questa convergenza, se non *in limine litis*, non la state cercando, e questo voto favorevole non lo cercate e forse neppure lo volete. E nel ribadirle che noi siamo ancora pronti a fare una riforma seria non contro i giudici ma per gli interessi di tutti i cittadini, attenderemo che nel prosieguo della legislatura, se tale prosieguo ci sarà, i segnali siano ben più chiari da parte del Governo e condivisibili, per poter così sostenere i suoi provvedimenti.

Alcune valutazioni, però, si fanno indipendentemente dalla relazione, perché tutti noi siamo spettatori e conoscitori del sistema.

ma quello è uno strumento della riforma strutturale, non è la riforma strutturale. La riforma strutturale annunciata e condivisa dal Ministro nel 2008 prevedeva la riorganizzazione degli uffici, strumento importante, e di quella non si è avuta più traccia. Nel 2008 il signor Ministro era d'accordo alla soluzione prospettata, materia di approfondimento, anche se già approfondita da almeno vent'anni e parzialmente sperimentata da alcuni uffici, come l'istituzione dell'ufficio per il processo; il Ministro era d'accordo, poi non se ne è più parlato. Una delle lacune più gravi che si avvertono - veramente tra le più gravi, e le conseguenze le conosceremo drammaticamente più avanti si andrà nel tempo - è che nel comparto giustizia non si assume dai primi anni Novanta il personale amministrativo sta invecchiando: è arrivato a una media di età di 55 anni. Non c'è l'ingresso dei giovani. Ogni anno vanno in pensione 900 dipendenti e non c'è *turn over*. La crisi che si sta verificando all'assenza del passaggio di conoscenze e di esperienze che prima caratterizzava gli uffici pubblici. Si impoveriscono, ed invecchiano naturalmente,

ai giovani che un domani verranno. Ma si può assistere a questo depauperamento? L'ufficio per il processo, così come da noi disegnato e condiviso dal Ministro,

alla Camera, in Commissione giustizia, che quel disegno di legge da noi presentato e da me coltivato aveva la copertura finanziaria e prevedeva la riqualificazione del personale e l'assunzione di 2.800 cancellieri. Non se ne è fatto nulla, è stato abbandonato. Si assiste allora alla mancanza di visioni strategiche. Questa era la legislatura in cui si poteva fare il discorso della geografia giudiziaria: le legislature lunghe consentono di farlo;

formulate nel corso del tempo. Infine, vorrei esprimere un giudizio complessivo. Sono rimasto sconcertato per aver assistito ieri sera ad un dibattito televisivo in cui il Ministro della giustizia faceva l'avvocato.

e quando noi insistemmo pregandolo di non dimettersi disse: «Voglio parlare dell'indagine che mi riguarda e fin quando sono Ministro non lo posso fare». Ora invece abbiamo un Ministro che va nelle trasmissioni televisive a fare l'avvocato, accusando la magistratura ed altri. Sobrietà! Anche lo stile e gli strumenti di intervento fanno parte di un bilancio,

Signor Presidente, colleghi, per motivare il voto contrario alla proposta di risoluzione della maggioranza che approva la relazione del Ministro mi collego all'*incipit* del collega Li Gotti. La frase finale del Guardasigilli ieri in quest'Aula attesta e dichiara la sua sconfitta. Mi riferisco all'ammissione che il 2010, l'anno in cui è stata annunciata la grande riforma strutturale della giustizia, è passato invano scandito, invece, da una serie di interventi interventi tampone tutti finalizzati a gestire le emergenze che derivano al Ministro ed al relativo Governo dalle precarie condizioni politico-istituzionali del Capo del Governo. infatti, dovessimo rintracciare il filo conduttore dell'iniziativa legislativa di questo Dicastero, troveremmo il tema del legittimo impedimento, il tema del processo breve, vedremmo l'opera attorno al lodo costituzionale e, e, *dulcis in fundo,* il grande tema delle intercettazioni: a leggere le cronache di questi giorni, si capisce la preoccupazione e l'impegno del Governo e della maggioranza attorno al tema delle intercettazioni! l'idea di una grande riforma che affronti il nodo strutturale della giustizia, della relazione tra i poteri, degli equilibri tra i poteri dello Stato in una

tipica di un Governo caratterizzato da grandi annunci di riforme cui non seguono fatti concreti, trattandosi di un Governo precario che vive una condizione di manifesta forza parlamentare ma di debolezza politica intrinseca. anche per le questioni più specifiche, signor Sottosegretario, ho apprezzato il tono, ho letto la volontà di allargare l'area di consenso in un momento così delicato politicamente proprio attorno al tema della giustizia. In tal non sono censurabili alcune indicazioni, come quelle date dal collega Li Gotti, sulla opportunità che il Ministro non interferisca nei procedimenti giudiziari con posizioni di parte. Egli ha un ruolo di garanzia straordinario e deve mantenere questa sobrietà. Ma anche attorno alle questioni più concrete, come il tema della durata irragionevole dei processi, non avete affrontato il problema con un provvedimento relativo alla procedura, all'organizzazione dei mezzi,

Per non parlare poi delle carenze di organico della polizia penitenziaria o di quella ancor più grave della magistratura nelle aree più difficili del Paese. Le posso citare le carenze drammatiche di organico nella Regione Sicilia, dove il tema del contrasto alla criminalità organizzata, ma anche della normale amministrazione della giustizia, rappresenta un diritto fondamentale. Il Ministro, che dovrebbe ben conoscere le

un'opera di razionalizzazione che consentirebbe di impiegare meglio uomini e mezzi e invece, per non urtare suscettibilità campanilistiche, non si mette mano alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Parliamo poi dei grandi vanti

apprezzo che si sia invertita la tendenza ma certo ieri era sbilanciata, signor Sottosegretario. Il Ministro ha sfuggito però i temi strutturali e fondamentali per concentrarsi su temi marginali sui quali poteva rivendicare qualche successo, facendo dimenticare carenze di iniziative

nel rivendicare a questo Esecutivo i successi nella lotta alla mafia. È vero, ma è un merito che va molto condiviso, per la gran parte con i magistrati e le forze di polizia, quegli stessi magistrati che spesso sono coloro che ottengono questi risultati e poi vengono criticati pesantemente dall'Esecutivo quando qualche indagine intacca la serenità e l'equilibrio di questo Governo. Per rivendicare i meriti ed ascriverseli occorre considerare con equilibrio la propria parte e non dimenticare chi fa il proprio lavoro e rischia in prima linea sul terreno durissimo del contrasto alla criminalità organizzata. al Presidente del Consiglio quando ancora, a settembre, votammo la fiducia al suo Governo (poi non l'abbiamo più fatto), fidandoci di alcune prospettive di riforma che aveva annunciato: gli spiegammo però che sulla giustizia, se le prospettive d'intervento erano quelle annunciate attorno a modifiche anche costituzionali che potevano ledere l'indipendenza e l'autonomia della magistratura o che avessero un carattere punitivo confronti dei magistrati, ci avrebbe trovato duramente contrari, e glielo confermo. Anche questo tentativo, evocato più volte, di mettere mano di legge costituzionale con interventi parcellizzati che abbiano come obiettivo vero quello di ridurre la capacità di controllo di legalità affidata alla magistratura è una scelta inaccettabile. Siamo disponibili - e l'abbiamo evidenziato nella nostra proposta di risoluzione - ad un confronto serio che affronti complessivamente la riscrittura di questo capitolo della Carta costituzionale e riveda complessivamente in modo aggiornato il sistema di relazione tra i poteri dentro il solco rigidissimo della separazione, in cui rimane fermo il principio dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. Per concludere, se il Ministro fosse meno impegnato a tamponare le emergenze (e lui da efficiente ed obbediente esecutore delle indicazioni collegiali o del leader del Governo deve ottemperare) e avesse più spazio

sono abbastanza vicini, forse sarebbe utile che il Ministero, per come è concepita oggi la sua azione, direttamente si trasferisse a Palazzo Grazioli, così ci sarebbe una costanza di impegno a tutela del vero bene che il Governo protegge, che è un bene costituzionale: il Presidente del Consiglio dei ministri. ministri. Per l'intero tempo del suo impegno, il Governo oggi è concentrato su questa attività. Palazzo Grazioli ormai è una sede istituzionale; tranne le ore notturne non opportune, può essere una buona sede per il nuovo Ministero della giustizia.

ma devo dirle con altrettanta sincerità e franchezza che siamo rimasti molto delusi dalla relazione del Ministro della giustizia, soprattutto se la confrontiamo con quella dell'anno precedente, in cui il ministro Alfano aveva esordito dicendo (cito testualmente) che «il 2010 passerà alla storia come l'anno della compiuta riforma ordinaria e costituzionale del sistema giudiziario». In realtà, tutto ciò non è avvenuto credo sia obiettivamente ingeneroso e forse anche infantile sostenere la tesi che le riforme che sono in Parlamento (mi riferisco a quelle ordinarie, che sono le uniche serie che si sarebbero dovute fare, che si dovevano fare e che si devono fare) che si devono fare) non possono andare avanti per le cosiddette tensioni politiche. Mi sembra una giustificazione infantile e poco riguardosa per il dibattito politico su un tema così delicato, complesso ed importante come quello della giustizia, che riguarda milioni di cittadini italiani e innanzi tutto il sistema economico e sociale del nostro Paese.

intenzionalmente sotto tono per cercare di sgattaiolare in Parlamento rispetto alla triste contingenza di ciò che da giorni siamo costretti a leggere sui giornali;

ai colleghi senatori che rivolgono le spalle alla Presidenza di smettere di chiacchierare e possibilmente di allontanarsi dall'Aula se non intendono ascoltare l'intervento del

leggere, anche in maniera demotivata, il compitino dell'ufficio statistica del Ministero della giustizia non credo sia un modo opportuno di affrontare il tema delle riforme,

non si sono mai sottratti ad un confronto di merito su tali questioni) ma quando siamo passati dall'esame dei princìpi alla scrittura delle norme da applicare ai casi concreti, ci siamo trovati di fronte a vere e proprie aberrazioni dal punto di vista giuridico. Cito due casi per tutti:

cosa dovrebbe dirci il Ministro della giustizia a fronte del fatto che il Presidente del Consiglio ritiene di essere un perseguitato politico sempre e comunque da parte della magistratura italiana?

dell'ex presidente brasiliano Lula, il quale ha negato l'estradizione ad un terrorista come Battisti affermando che nel nostro Paese non sono salvaguardati i diritti fondamentali della persona umana, a cominciare

nega l'estradizione, perché ritiene che in Italia i magistrati non facciano il loro dovere con imparzialità? Questo è il punto. Comprendo dunque ministro Alfano, e sono umanamente solidale con lui nel momento in cui non viene in Aula e fa una relazioncina che ci sembra un po' - senza offesa - il conto della serva su

il fallimento di una politica di riforme tutta orientata a risolvere singole, specifiche questioni giudiziarie e processuali e non i problemi dei cittadini italiani. Per questo, noi valutiamo negativamente la relazione del Ministro, perché condensa una politica giudiziaria fallimentare, al di là di piccoli interventi e di specifiche questioni sulle quali non abbiamo alcuna difficoltà

riguardano le confische e l'aggressione ai patrimoni mafiosi e, perché no, anche con riferimento ad altre questioni che hanno riguardato l'abbreviazione del rito civile; resta però

in una Cinquecento il motore di una Ferrari: se non funziona la macchina non può funzionare il motore. Si semplifica una parte del rito civile, ma si mantiene la complessità e la molteplicità dei riti

l'imparzialità dell'attività del magistrato, costretto ad avvalersi sul territorio di quelle scarse risorse umane e strumentali per gestire delle circoscrizioni giudiziarie piccole, che lo costringono anche un contatto quotidiano

la moltiplicazione e l'insostenibilità del numero delle circoscrizioni giudiziarie nel nostro Paese determina un problema di disorganizzazione, di polverizzazione delle risorse e rende impossibile coprire gli organici, perché

si voglia scherzare. Veramente il ministro Alfano ritiene che i problemi della giustizia si affrontino e si risolvano con una riforma costituzionale che, nella migliore delle ipotesi e se dovesse veramente vedere la luce, dopo un ampio e approfondito dibattito parlamentare, comincerà a produrre i suoi effetti fra tre anni? In questi tre anni cosa facciamo? Della riforma del processo penale che è pendente in Parlamento cosa facciamo? Della riforma della professione forense, che con grande difficoltà questa Aula ha licenziato, perché anche lì i pasticci non mancano, cosa facciamo? Quegli interventi strutturali, che si dovrebbero fare con legge ordinaria e che sono tanti, possiamo non farli perché vi sono una serie di questioni, di contraddizioni e di tempi parlamentari che se utilizzati sacrificherebbero altri provvedimenti che forse, in tema di giustizia, bisogna con urgenza portare avanti? Sul tema della riforma costituzionale le vogliamo dire con grande chiarezza, signor Sottosegretario, che la riforma che dobbiamo fare è quella di applicare il principio dell'unità e dell'unicità della giurisdizione e degli organi di autogoverno. autogoverno. Non possiamo avere quattro magistrati che giudicano lo stesso fatto da un punto di vista giuridico diverso, perché tutto questo ha determinato in questo Paese l'irragionevole durata dei processi, il conflitto di giudicati e l'incertezza del diritto, altro che separazione delle carriere, altro che dibattiti

questi manifesti ideologici che non servono a niente e che hanno reso e continuano a rendere la giustizia un terreno di confronto e di scontro strumentale, ma non per risolvere le questioni cui i cittadini italiani sono particolarmente interessati. Su questo tema, mi consenta di dire che forse il Presidente del Consiglio dovrebbe andare dai magistrati alle questioni di merito che sono oggetto di altro apprezzamento - per dare anche un messaggio di serenità al nostro Paese e ai cittadini italiani;

ha definito, ma perché non è condizionabile dall'ultima ragazzina che entra a casa sua; per dire che è sereno perché la sua credibilità internazionale e di questo Paese, in un momento di crisi economica e sociale, non è messa in discussione.

era inevitabile che questo dibattito sullo stato della giustizia avesse questo tipo di risvolto.

maniera. Noi non siamo così ingenerosi nel dare il giudizio sull'attività del Ministero parlando di riforme fallimentari. Probabilmente ogni cosa può essere vista con lenti diversi; ognuno ha occhiali diversi:

Se vogliamo essere onesti, l'unico dato che emerge è che l'accumulo di arretrato è arrivato ai livelli massimi fino al 2009 e solo nel 2010 abbiamo visto uno smaltimento di circa il 5 per cento di pratiche rimaste nei secoli nella storia inevase. Dovremmo quantomeno riconoscere che la giustizia ha avuto uno scatto d'orgoglio. È dipeso da cosa? Sarà dipeso un po' da tutto e anche da qualche piccola riforma portata a casa. il nostro lavoro si è concentrato sul migliorare l'efficienza della macchina degli uffici per eliminare la lentezza burocratica della giustizia e questi sono gli unici due filoni

invece che presso un carcere mandamentale o circondariale, la propria pena. Un'altra verità assoluta è che viviamo momenti di ristrettezza in ogni campo, dall'ambiente alla giustizia - ogni tanto parliamo di difesa - alla scuola e alla ricerca. Si recrimina che non vi siano risorse sufficienti.

quando si è parlato molto in quest'Aula di intercettazioni. Ricordo che la procura d'Italia che ha speso minori risorse in intercettazioni (ha speso un decimo rispetto alla media nazionale) è quella che ha ottenuto maggiori successi sotto il profilo

28 superlatitanti su 30 nel giro di due anni. Reputo questo un risultato da riconoscere all'amministrazione della giustizia, ai magistrati che hanno compiuto il loro lavoro, agli agenti di polizia, a tutte le strutture e anche ai due Ministeri che hanno dato un certo impulso e hanno tenuto la regia della situazione.

dovrebbe fare un piccolo esame di coscienza e riconoscere che il dato oggettivo non è quello che istintivamente e ideologicamente si vorrebbe far passare. Abbiamo altrettanto apprezzato una cosa apparentemente normale. Infatti, la realizzazione di progetti

house*, cioè con gli uffici tecnici e le strutture che si hanno a disposizione. Finalmente si valorizzano le risorse interne perché ormai la pubblica amministrazione è

mai come oggi è il caso che proprio dai livelli politici arrivi anche un segnale all'ordine della magistratura. In quest'Aula ci sono tanti magistrati. Bisogna far capire una cosa banale: la giustizia è un servizio la giustizia è un servizio per i cittadini e i giudici non sono dei principi nel palazzo da doversi ossequiare e riverire, bensì servitori

esprime una classe politica che vorrebbe fare quattro regole e vederle rispettate e non stravolte da parte di una classe di magistrati che ormai si è arroccata e pensa di poter dettare legge per questo Paese.

Ora lasciamo che le indagini facciano il proprio corso, ma non si era mai visto un capo d'imputazione di concussione

un'imputazione per sfruttamento della prostituzione quando la presunta vittima ha dichiarato di non aver mai avuto rapporti con il soggetto imputato. Signor Sottosegretario, bisogna riportare nel giusto binario chi oggi tende, spesso e volentieri, a deragliare.

Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, è francamente difficile discutere su di una relazione, quale quella di ieri del Ministro della giustizia, così dimessa, inconcludente e priva di prospettive; in effetti, più idonea ad un clima da basso o forse fine impero. Così diversa dalle dichiarazioni e dai proclami roboanti, in materia di giustizia, del presidente del Consiglio Berlusconi e del suo Ministro Guardasigilli. Essi ci avevano abituati, anche in quest'Aula, a promesse di grandi interventi, a promesse di una grande, grande, grande, sei volte grande, riforma della giustizia. E invece ora sembra tutto scomparso. Anzi, peggio: dopo quasi tre anni di questo Governo, dopo otto degli ultimi dieci anni governati dal premier Berlusconi, ci si viene letteralmente a dire che i progetti del Governo sono stati e sono spesso ostacolati fisiologicamente dall'estrema complessità delle questioni da affrontare, dalle difficoltà economiche e dallo schema di bilancio troppo rigido e vetusto, oltre che, patologicamente, dall'eccessiva polemica politica e da resistenze anche interne al sistema giudiziario. Secondo il Ministro, però, molti e rilevanti sarebbero stati i risultati conseguiti. Imponente, per il Ministro, sarebbe stato l'impegno del Governo. Ma noi ci chiediamo: dove? Quando? Su che cosa? Certo, se il Ministro Guardasigilli si riferisce al suo impegno, anche personale, nel cercare di risolvere i problemi individuali e processuali del Premier e della cricca, ha ragione. Ha perfettamente ragione. Va dato atto a lui e ai "consigliori" del Premier di aver provato a fare di tutto, ma proprio di tutto, per sottrarre Berlusconi e la cricca a indagini e processi. Fatica che va riconosciuta, per loro certamente encomiabile, bloccata però, e per buona sorte, da una opposizione democratica e da una Corte costituzionale ligie ai principi di legalità e di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, come sanciti dalla nostra Costituzione. A dire il vero, tanto impegno e tanti sforzi del Governo avrebbero dovuto tendere ad obiettivi diversi, quelli che realmente interessano e toccano molto da vicino il cittadino e la collettività, i problemi ormai arcinoti attinenti alla lentezza dei processi (civili, penali e anche amministrativi), alla efficienza della macchina giudiziaria e alla effettività delle decisioni giudiziarie. La nostra critica severa, come Partito Democratico, nei confronti del Ministro non è pregiudiziale né ideologica, perché ad esempio in tema di lotta alla mafia abbiamo decisamente e fortemente contribuito all'approvazione di norme efficaci. parlo di una nostra opposizione non pregiudiziale né ideologica perché fin dall'inizio di questa legislatura, ormai circa tre anni fa, come Partito Democratico le abbiamo presentato tutta una serie di proposte di legge, concrete e specifiche, alcune delle quali anche ieri ed oggi abbiamo illustrato e comunque elencato nella nostra dettagliatissima proposta che dovrebbe essere letta accuratamente e che costituisce la *summa* di un nuovo nostro programma alternativo di governo del sistema giustizia. E lo abbiamo fatto perché siamo realmente convinti della gravità della situazione, dello stato fallimentare in cui versa la nostra macchina della giustizia e dell'assenza totale di proposte del Governo e della maggioranza di destra attuali. Ma da parte vostra nessuna risposta: peggio che orecchie da mercante! Da parte vostra, antenne ritte solo per norme e provvedimenti a tutela della cricca, volte a rendere sempre più difficili le indagini, norme come quelle che avete presentato al Parlamento un paio d'anni fa e ieri riproposto in tema di intercettazioni. Vecchie norme bocciate già dalle istituzioni e dalla opinione pubblica, che potrei sintetizzare dicendo che ancora una volta volete mettere il bavaglio alla stampa e le manette a poliziotti, carabinieri e magistrati, terrorizzati dal rischio che si vengano ad accertare e conoscere fatti di corruzione, malaffare o da postribolo. Relazione dimessa, ho detto, ma forse sarebbe più appropriato definirla penosa o pietosa, in presenza di una enfatizzazione dell'attività del Governo che lei, signor Ministro, francamente ha provato ad operare, pur con poca convinzione e tra critiche pur sommessamente formulate da senatori della sua stessa maggioranza, ad esempio, in tema di processo civile, di media conciliazione o di mancata riforma del cosiddetto tribunale della famiglia a tutela soprattutto dei minori. E non c'è da aggiungere altro sulla tutela dei minori, anche se mi verrebbe da chiedere: ma che fine ha fatto il tanto decantato disegno di legge del ministro Carfagna sulla lotta alla prostituzione? Tanto strombazzato e ora *desaparecido*, nascosto nei cassetti polverosi della 1a e della 2a Commissione? La disfatta del sistema giustizia è sotto gli occhi di tutti. Non serve al Ministro, giocherellare coi pochi numeri che ha: piegare le statistiche, ad esempio, sul numero dei processi civili ai suoi *desiderata* se idee per davvero non ne ha, se idee non ne avete. ha dedicato circa 400 righe della sua relazione al tentativo di magnificare il nulla della proposta di Governo, riservando nelle conclusioni una decina di righe al riconoscimento della mancata, da parte vostra, riforma della giustizia ovviamente per colpa dell'evoluzione del quadro politico, delle tensioni di fine 2010, come se tensioni e modifiche del quadro politico non fossero un problema tutto interno a voi ed alla vostra maggioranza ormai incapace di governare. E così, in poche righe il Ministro finisce per bofonchiare richiami a non si sa quale riforma o innovazione del sistema, privi di ogni aggancio con la realtà e con le necessità quotidiane, salvo però ricordarsi di ribadire quanto preme davvero al Premier, cioè che il regime delle intercettazioni telefoniche sia assolutamente modificato. Ma dove vive questo Ministro Guardasigilli e dove vivono i suoi "consigliori" e preparatori di bozze? Pensano forse che le esigenze della giustizia siano quelle che emergono dalla villa di Arcore o dalle telefonate di prostitute e prosseneti? Ci vuole altro, signori del Governo! Stupefacente poi è il modo in cui con la relazione di ieri il Ministro ha menato il can per l'aia, raccontandoci dei suoi rapporti internazionali e della sua partecipazione ad un'Assemblea dell'ONU come spettatore. Ma noi invece che sentir parlare di un trattato di estradizione con la Cina, alla quale i peggiori criminali cinesi non potranno comunque mai essere dati, avremmo preferito sentire di come il Governo e la maggioranza intendano giuridicamente tutelare le nostre imprese, le nostre industrie e i nostri lavoratori dalla aggressione economica e finanziaria del colosso asiatico. signor Ministro si è trovato all'Assemblea dell'ONU, avremmo preferito sentire come il Governo e la maggioranza intendano dare concreta attuazione alle norme in materia di lotta alla corruzione originate dalla Convenzione ONU anticorruzione, approvate dal Parlamento con il disegno di legge del Partito Democratico. In conclusione, voglio utilizzare nella sostanza le parole del Ministro per ribadire quale sia il problema maggiore in tema di giustizia. Una preoccupante carenza di disegno strategico ed una sorta di anarchia decisionale ed operativa, che il Ministro cerca di attribuire al solo passato come se voi, negli ultimi 10 anni, foste stati sulla Luna o su Andromeda. Ecco, signor Sottosegretario, signori del Governo, questo è il problema: carenza di disegno strategico ed anarchia decisionale ed operativa. Ed allora, invece di correre al capezzale processuale di un Premier decadente sotto ogni profilo, si ricordi di quanto stabilito dall'articolo 110 della nostra Costituzione sul ruolo del Ministro della giustizia, che non è quello di segretario *sui generis* del Premier. soccorra, vada davvero al capezzale di questo nostro derelitto e decadente sistema giustizia; se ne ha e ne avete la capacità e la forza politica intervenite davvero. In caso contrario non vi resta che passare la mano.

Signor Presidente, colleghi senatori, signor Sottosegretario, signori del Governo, in un Paese normale ciò che il ministro Alfano ha comunicato ieri al Parlamento sarebbe stata la notizia del giorno. Tutte le forze politiche se ne sarebbero rallegrate senza distinzione, gli operatori della giustizia avrebbero condiviso con il Governo un meritato orgoglio e le forze produttive sarebbero corse a complimentarsi. Per la prima volta dopo decenni, infatti, il numero dei processi civili pendenti ha avuto un forte decremento, segnando un'inversione rispetto ad un *trend* disastroso. Per la prima volta dopo decenni, grazie al combinato disposto di riforme incisive e di una coraggiosa opera di razionalizzazione, possiamo sperare che venga recisa la zavorra che frena gli investimenti e tarpa le ali alla nostra economia, che soffoca la voglia di intraprendere, che allontana dall'Italia imprese e capitali produttivi. Senza contare che importanti misure destinate a deflazionare ulteriormente il contenzioso civile non sono ancora entrate a regime e, dunque, devono ancora produrre i loro effetti. Si tratta di una notizia importante, ma non è la sola che si può desumere dalla relazione, per chi la legge con occhi giusti e non con un insopportabile pregiudizio. Il Ministro della giustizia ha dato conto al Parlamento di un anno di silenziosa operosità. Mentre il Paese era stordito dal frastuono delle polemiche, dal ronzio dei controcanti, il Governo, con il convinto sostegno e il contributo di questa maggioranza, ha prodotto innovazioni sul piano normativo e passi da gigante in termini di modernizzazione dei procedimenti e di razionalizzazione degli uffici. Mentre nelle aule di giustizia nei salotti televisivi si alternavano sedicenti pentiti e nuovi "oracoli" - ieri a Firenze è andata in scena una nuova puntata della *fiction* - il centrodestra di maggioranza e di Governo, giocando in squadra con le forze dell'ordine e l'autorità giudiziaria, sferrava, in termini di leggi ed interventi operativi, la più incisiva azione di contrasto alla criminalità organizzata di cui si ha memoria nella storia dell'Italia repubblicana, giungendo tra l'altro a sottoporre il più alto numero di boss mafiosi al regime del 41-*bis* dall'anno della sua introduzione. Mentre le opposizioni rifiutavano di fare i conti con le ricadute della crisi, imputando al Governo l'esigenza di tenere a posto i conti del Paese, il Governo, nonostante quella stessa crisi e grazie anche alla razionalizzazione della spesa, ha nominato centinaia di nuovi magistrati e per altrettanti ha bandito concorsi, facendosi altresì carico di rimuovere con misure straordinarie gli impedimenti per la copertura di uffici vacanti e sedi disagiate. Infine - e mi preme sottolineare questo dato tra i tanti che il ministro Alfano ci ha fornito - il Governo ha affrontato l'emergenza carceraria con una energia e una determinazione che mai il sistema penitenziario italiano aveva conosciuto prima d'ora. A cominciare dal massiccio apporto di risorse umane previsto per la polizia penitenziaria, dalle nuove strutture edilizie previste nel piano carceri, e dal complesso di interventi normativi per affrontare alla radice il dramma del sovraffollamento. Questa è la politica del Governo in tema di giustizia, queste le emergenze di cui la maggioranza si sta facendo carico. C'è però un'altra emergenza, che molti di voi vorrebbero non vedere o vedere in modo distorto, nonostante da 20 anni a questa parte gli eventi si siano ciclicamente incaricati di renderla drammaticamente evidente. È un'emergenza per la cui soluzione il Paese si aspetta non solo la determinazione della maggioranza, ma anche il contributo di quanti non vorranno consegnare alle future generazioni una democrazia a sovranità limitata. All'attuale maggioranza, che da 17 anni patisce il tentativo di rovesciamento della volontà dei suoi elettori per via giudiziaria; e all'attuale opposizione, che appena tre anni fa ha visto concludersi la propria esperienza di Governo non solo per conflittualità interna, ma anche e soprattutto per l'incursione di una procura di provincia dichiaratamente incompetente a indagare, e per i bombardamenti di un pubblico ministero, ora eurodeputato, su cui pende una richiesta di rinvio a giudizio per la disinvoltura con cui ha maneggiato i dati telefonici dei parlamentari; a tutti noi, al di sopra e al di là dei polveroni contingenti, spetta l'onere di ricucire quel drammatico strappo tra giustizia e politica provocato nel nostro Paese da una frettolosa ed emotiva rottura dell'equilibrio costituzionale che si è consumata con la revisione dell'articolo 68 della Costituzione sull'onda di tangentopoli. Se iniziano a parlarne anche eminenti magistrati (cito fra tutti il presidente della corte d'appello di Bari Vito Marino Caferra), se ne parlano anche autorevoli politici della sinistra (come Giuliano Pisapia), forse il tempo è maturo perché i rappresentanti del popolo si assumano le proprie responsabilità, anche e soprattutto in un momento come questo. Vede, collega senatrice Finocchiaro, glielo dico con la stessa chiara determinazione che ha usato lei: in un momento nel quale si formulano richieste e ipotesi di reato infamanti, chiedere giustizia, chiedere chiarezza, soprattutto, è doveroso, ma per farlo bisogna innanzitutto occuparsi della condizione del nostro Stato di diritto,

se si mettono da parte le strumentalizzazioni e ci si rende impermeabili alle sirene del giustizialismo e alla tentazione di imboccare improvvide scorciatoie, non sfuggirà a nessuno, nemmeno a tanti colleghi dell'opposizione, la deformazione che negli ultimi anni ha cambiato i connotati del nostro Stato di diritto. L'accrescersi del potere "creativo" della giurisprudenza ha infatti infranto il già fragile legame che univa il potere giudiziario al circuito della sovranità del popolo, ovvero l'esclusiva soggezione del magistrato alla legge dello Stato. Con il tempo questo meccanismo ha trasformato l'ordine giudiziario in un potere di fatto irresponsabile. In campo penale, gli spazi di discrezionalità sono diventati arbitrio, e la spettacolarizzazione della giustizia unita all'insopportabile lentezza dei processi ha fatto sì che il contraddittorio tra le parti, la formazione della prova e il giudizio finale fossero schiacciati sotto il peso dei fuochi di artificio preliminari, dell'applicazione disinvolta di misure preventive, dell'abuso di strumenti di indagine altamente invasivi della sfera intima delle persone; dal Gruppo PdL)*, delle accuse unilaterali, degli indizi e dei meri sospetti tramutati in condanna preventiva. Non è più importante né il processo, né la sentenza; la cosa importante è l'effetto che si produce prima. Con questo sistema sono stati fatti fuori assessori regionali di una parte e dell'altra, dei cui processi si è persa ogni traccia; si sono abbattuti Ministri mai neppure iscritti nel registro degli indagati. Con questo sistema si vorrebbero ora, e per l'ennesima volta, instaurare nuovi cicli politici che alla democrazia del popolo sostituiscano la volontà di un'*élite* di ottimati. Colleghi delle opposizioni vecchie e nuove, non illudetevi che l'uso politico della giustizia possa essere uno strumento di cui avvantaggiarvi oggi a danno del centrodestra senza pagarne lo scotto in futuro. Senza scomodare Pietro Nenni e il suo celebre ammonimento sul più puro che ti epura, basta osservare quale conflitto intestino stia dilaniando il partito giustizialista per eccellenza. Assumiamoci tutte le responsabilità,

(proprio nei momenti più difficili si vede la qualità delle classi politiche). E sulla scia dei nostri Padri costituenti ripristiniamo ora ripristiniamo ora l'equilibrio spezzato, per restituire al popolo la sua sovranità e alla giustizia la sua sacrosanta autonomia,

Esso prevede che l'articolo 68 della Costituzione torni ad assomigliare a ciò che era in origine, consentendo alla Camera di appartenenza di disporre entro un certo termine la sospensione di un eventuale processo a carico dei rappresentanti del popolo, rinviandone il decorso al momento in cui sia cessato il mandato democratico *(Applausi dal Gruppo* *PdL)*. Ripartiamo da qui, senza cedimenti al giustizialismo. Sarebbe il modo migliore affinché la richiesta di chiarezza la richiesta di chiarezza non sia offuscata dalla strumentalità, per onorare quel patto costituente al cui rispetto ogni giorno ci sentiamo richiamare. *(Applausi

tabù in tutto questo dibattito che invece noi radicali, non da oggi e non da soli, portiamo avanti da tanto tempo

oggi un'amnistia strisciante, al di là di qualunque controllo parlamentare, che va sotto il nome di prescrizione, e dai dati ufficiali del Ministero le prescrizioni ogni

proprio per evitare di divenire tutti antipopolari, senza volerlo e senza saperlo, divenendolo di fatto nella realtà e nella gestione di ogni giorno. Sono milioni i cittadini italiani che aspettano giustizia.

Grazie

la vicenda dei rifiuti nella Regione Campania ha rappresentato un'emergenza sino dal 1994 ed è stata oggetto di provvedimenti straordinari che hanno reso necessaria l'individuazione

Questa legislatura è iniziata con l'esame del decreto-legge n. 90 del 2008, e successivamente ha visto altri provvedimenti con i quali è stata affrontata con vigore e determinazione un'emergenza giunta a livello di criticità nazionale e che, occorre ricordarlo, ha offerto un'immagine negativa del nostro Paese nel contesto europeo e internazionale. L'impegno del Governo, che per una fase è stato diretto anche nell'operatività della gestione dei siti e delle modalità di smaltimento, nell'individuazione degli impianti e delle loro modalità di realizzazione, ha avuto nel corso del 2009 il subentro dalla responsabilità nazionale a quella degli enti territoriali: enti che, come deve essere e come avviene nel resto d'Italia, debbono istituzionalmente occuparsi della gestione dei servizi pubblici locali e, in specie, del ciclo dei rifiuti. Se da un lato non può essere negato il miglioramento strutturale della situazione, l'attivazione di impianti, la crescita della raccolta differenziata e anche la progressiva assunzioni di responsabilità da parte degli enti locali che nel passato avevano fallito, dobbiamo registrare ancora oggi ritardi e difficoltà. e difficoltà. Se non era corretto, circa due anni fa, accomunare nel ritardo e nell'emergenza campana tutti i Comuni della Campania, non possiamo oggi oggettivamente negare che in molte realtà territoriali

se è necessario, come infatti è, accompagnare la progressiva realizzazione di sistemi di gestione dei rifiuti in Campania verso una consolidata e duratura normalità non si può, come nel dibattito in Commissione si è tentato di fare, affermare che nulla è cambiato e che la situazione in atto sia la medesima di quella della primavera del 2008. Per questa ragione il presente decreto non sottrae, come avvenne nel 2008, la diretta competenza statale a quella di Regione, Province e Comuni e non avoca alla responsabilità dello Stato la gestione di un'emergenza frutto del fallimento di un sistema territoriale, ma conferisce poteri e deroghe alla Regione e ai Comuni campani, nella logica di un aiuto significativo per procedere, secondo una direzione impostata dal sottosegretario di Stato Bertolaso, ad un lavoro già avviato con successo in molte realtà provinciali ed oggi da completare anche nella città di Napoli e in altri territori che ancora sono in difficoltà. Occorre quindi prorogare alcune norme derogatorie. Occorre prevedere ancora alcune modalità non ordinarie per l'individuazione di altri siti di smaltimento,

Serve, questo decreto, che non banalizza i problemi che ci sono, ma pone, a differenza del passato, la centralità della Regione Campania, delle sue Province e Comuni, e non la surroga o la sostituzione di queste istituzioni. Sono certo che il dibattito approfondirà gli specifici contenuti del provvedimento. La maggioranza e lo stesso Governo si sono presentati favorevoli alle proposte di miglioramento ed al confronto. Il dibattito e il confronto continuano oggi nell'Aula parlamentare del Senato anche su un nuovo emendamento, presentato dal relatore d'intesa con il Governo, per accogliere sostanzialmente un emendamento utile presentato dall'opposizione su un contenuto già oggetto di un ordine del giorno, di cui primo firmatario è il collega De Luca, sull'utilizzo prioritario delle cave abbandonate e dismesse come potenziali siti di stoccaggio dei rifiuti. rifiuti. In conclusione, annuncio che sono stati presentati alcuni emendamenti per dare conto a rilievi tecnici della Commissione bilancio.

*(PD)*. Signor Presidente, signora Ministro, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, su questo argomento bisogna resistere alla tentazione della strumentalità, lasciando prevalere obiettività ed onestà intellettuale. Non bisogna però tacere gli scenari di contesto in cui il problema si inquadra, e cioè l'interesse della malavita organizzata e le sue infiltrazioni nella gestione dei rifiuti, e perciò le innumerevoli discariche abusive, nel tempo disseminate sul territorio campano; l'accoglienza mai negata ai rifiuti industriali e tossici provenienti da altre Regioni, in particolare dal Nord Italia; le debolezze delle classi dirigenti locali; il ritardo culturale delle popolazioni nell'approccio con la risorsa rifiuti; i veti incrociati relativamente alle localizzazioni dei vari impianti del ciclo, persino da parte di esponenti della Chiesa cattolica locale; le divisioni che, per un lungo tempo, hanno caratterizzato oltre che il mondo politico anche quello scientifico, riguardo - ad esempio - le tecniche di smaltimento; l'inadeguatezza delle tecnologie prescelte per gli impianti di smaltimento programmati a seguito di una gara europea espletata nel 1998. Nel rileggere la storia tormentata dell'emergenza rifiuti in Campania ci si rende conto di quanto un tema, già di per se stesso difficile, divenga una matassa inestricabile, capace di compromettere - spero in modo non irreversibile, naturalmente - l'immagine di un territorio che, pure al proprio interno, detiene tante eccellenze ed è in grado di vantare per storia, per tradizioni di civiltà, valori ambientali diffusi, patrimonio paesaggistico, archeologico, architettonico, artistico e culturale. Non è il momento, né sarebbe opportuno farlo, di ripercorrere alcune tappe di questa lunga e dolorosa vicenda. Vorrei semplicemente sottolineare che la prima dichiarazione dello stato d'emergenza nel settore dei rifiuti, in Regione Campania, risale all'OPCM 11 febbraio 1994. Da quella data ai nostri giorni lo stato d'emergenza è stato via via riconfermato e altri nove commissari di Governo si sono avvicendati. Nel maggio 2008 il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, all'epoca e fino all'11 novembre 2010 anche capo della Protezione civile, assunse la delega all'emergenza rifiuti in Campania. Salto per brevità i passaggi intermedi che videro protagonista e poi dimissionario lo stesso dottor Bertolaso durante il Governo Prodi 2006-2008.

non vi era, d'altronde, alcuna consapevolezza negli amministratori locali del Mezzogiorno della gravità dei problemi, né la minima capacità di individuare le ricadute nefaste sui territori.

una comunità locale. Ebbene, i poteri straordinari venivano conferiti in parte al prefetto di Napoli, ma già all'epoca, in altra parte, e più ancora in seguito, al Presidente della Regione, cioè a chi nella funzione ordinaria di quell'ente aveva determinato l'emergenza. seguente. Ho fatto cenno all'istituzione, e non individualmente a chi, nel tempo, dal 1994 fino ai primi anni 2000 in poi, ne ha rappresentato il vertice: voglio dire che la Regione come soggetto istituzionale non è riuscita a governare il settore né attraverso poteri ordinari né con poteri straordinari. Cito un solo esempio: il il termovalorizzatore di Acerra, che fu previsto nell'originario piano di smaltimento definitivo dei rifiuti (1996: giunta regionale di centrodestra guidata dal presidente Rastrelli) e dalle successive elaborazioni sostanzialmente mantenuto, fu aggiudicato con gara del dicembre 1998. Una prima consegna delle aree avvenne il 23 gennaio 2003, cinque anni dopo; poi vi fu un'occupazione prolungata da parte dei manifestanti fino all'agosto 2004; l'aggiornamento del parere di compatibilità ambientale rilasciato nel 1999 fu acquisito dal commissario delegato nel febbraio 2005, circa un anno dopo la richiesta. precisazione: ho detto «fino ai primi anni 2000» perché dalla prima metà del 2004 in poi il presidente della Regione Campania, Antonio Bassolino, non ha più i poteri commissariali, che vengono posti in capo ad altri soggetti (il prefetto Catenacci e altri ancora). Dunque, siamo di fronte ad un fallimento complessivo delle istituzioni, a qualunque livello, locale, regionale e statale, in qualunque stagione da qualunque segno politico guidate, ed in presenza costante (solo negli ultimi tempi registriamo positive controtendenze) di una immaturità delle classi dirigenti locali e dei cittadini nella gestione dei rifiuti, nelle più elementari pratiche di raccolta differenziata, ai veti incrociati di gruppi organizzati, di forze politiche, di esponenti delle alte gerarchie ecclesiastiche rispetto a determinate ipotesi allocative. E non mi riferisco alle reazioni degli ultimi periodi, oggettivamente comprensibili quando non affidate alla violenza, ma ad episodi del passato, che hanno fortemente condizionato il tormentato *iter* di certi processi. Perciò, poi, mi risulta veramente difficile capire certe criminalizzazioni sommarie, l'individuazione di un capro espiatorio, l'addossamento delle responsabilità su di una o due persone, come se chi è poi subentrato negli stessi ruoli non avesse incontrato le medesime difficoltà. che lo stesso Presidente del Consiglio ha dovuto prendere atto talvolta della impossibilità di mantenere date, impegni, e che la Protezione civile, che in tante circostanze ha dato prova di sé, ha dovuto scontrarsi contro incrostazioni, mentalità particolari, particolari, resistenze non sempre motivate. È capitato e capita, signor Presidente, signora Ministro, che il sindaco di Napoli venga additata come la responsabile persino di quanto accade nei Comuni dell'*hinterland*, notoriamente esorbitanti della sua competenza, guidati da amministrazioni e sindaci di eguale o differente colore politico; come da altro colore politico è condotta da quasi due anni la Provincia di Napoli. Eppure quante volte anche in quest'Aula ho dovuto sentire ingiuriare il nome di Antonio Bassolino, di Rosa Russo Iervolino. Si è commesso un errore, un grave errore, perché non bisogna addossare le responsabilità in capo ad una persona, ma individuare nella risposta matura e consapevole delle classi dirigenti e

da due anni e mezzo c'è un Governo di centrodestra e ancora ci si attarda in polemiche inutili, esponendo talvolta oltremisura persone oneste e perbene, ponendo, seppure non intenzionalmente, a repentaglio la loro sicurezza personale e familiare e la loro incolumità fisica. Vorrei solo ricordare solo ricordare che questo è il secondo provvedimento che il Governo presenta, dopo il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, salvo poi la introduzione di alcune norme nel decreto Abruzzo, anche quelle relative al problema della normalizzazione dello stato di emergenza per i rifiuti in Campania. Accadde altrettanto durante il Governo Prodi: due decreti-legge riguardanti l'emergenza Campania, uno dei quali affidava al capo della Protezione civile, dottor Bertolaso, il compito di commissario di Governo. Come pure va detto che altre Regioni hanno attraversato e qualcuna ancora attraversa fasi emergenziali in tema di rifiuti, con il rischio sempre incombente che riaffiorino anche in modo eclatante: per esempio la Sicilia, la Calabria, la Puglia, il Lazio. Tornando al decreto-legge che il Senato è chiamato oggi a convertire in legge, sulle questioni di merito a nostro giudizio più rilevanti ci riserviamo, insieme con altri colleghi del Gruppo del di intervenire in sede di illustrazione degli ordini del giorno presentati e di dichiarazione di voto sui singoli emendamenti. Cito per tutti il tema della definizione delle competenze degli enti locali, anche al fine di accantonare taluni conflitti istituzionali in atto su pezzi di territorio

Quanto al sistema impositivo relativo all'esazione della TARSU, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e della TIA, la tassa integrata ambientale, riteniamo che sia assolutamente indispensabile lasciare ai comuni le competenze di raccolta dei rifiuti e di riscossione dei tributi e che altre ipotesi siano destabilizzanti, direi addirittura fuori dalla logica naturale delle cose, e ne risentirebbe oltretutto la qualità del servizio, la sua efficienza e naturalmente le conseguenze si abbatterebbero sull'utenza. È poi sostanzialmente poi sostanzialmente disatteso il principio della vicinanza territoriale tra impianti e luoghi di maggiore produzione dei rifiuti, che rappresentava un caposaldo del decreto Ronchi in piena sintonia con le direttive europee. Abbiamo tentato, pur nella consapevolezza da sempre sostenuta di prevedere meccanismi sanzionatori per le amministrazioni inadempienti, di introdurre una linea più equilibrata di fronte a tali fattispecie, meno affidata alla discrezionalità e dunque poggiata su presupposti e motivazioni meglio definiti, cosi ché non si determinino effetti dirompenti quando vi siano da parte delle amministrazioni comportamenti di inadempienza rispetto, per esempio, alla percentuale di raccolta differenziata. Proporremmo quindi di evitare effetti dirompenti e pericolosamente limitativi delle scelte del corpo elettorale locale e degli stessi principi democratici. È ben diversa dunque - e concludo, signora Presidente - l'idea che il Partito Democratico ha maturato e che ha responsabilmente esplicitato in un disegno di legge dei suoi Gruppi di Senato e Camera, presentato lo scorso novembre, illustrato anche al mondo dell'informazione, primo firmatario il senatore De Luca che certamente più tardi, in sede di dichiarazione di voto a nome del Gruppo PD, ne darà cenno.

pervenire alla definizione di norme semplici e chiare che favoriscano il ritorno alla normalità e stabilizzino l'ordinarietà.

il Senato della Repubblica nella imbarazzante condizione di provvedere alla conversione in legge, pochi mesi dopo avere ratificato -nel precedente provvedimento su analogo argomento - la fine della cosiddetta emergenza rifiuti in quella Regione. È innegabile che il Parlamento si sia trasformato (ed oggi ancora sia costretto da questo decreto-legge a trasformarsi) sia in un surrogato sia del Consiglio regionale della Campania, sia dei Consigli comunali e dei Consigli provinciali interessati, sia nel sostituto dei commissari succedutisi con inettitudine lungo questi ormai troppi anni. Ciò che inquieta ulteriormente in questo decreto-legge, anche con riferimento alle modifiche introdottevi nel passaggio alla Camera dei deputati, è l'impressione di una assoluta mancanza di strategia di sistema e di determinazione operativa. Non c'è, infatti, alcuna certezza di una inversione di rotta (nel senso di una consapevole assunzione di responsabilità politiche, amministrative e civiche) da parte delle istituzioni locali (regionali, provinciali e comunali). Non c'è, quindi, alcuna certezza né di tempi né di modi per garantire - da parte dello Stato - a quelle popolazioni che l'emergenza (che - anzi - non si vuole nemmeno più così definire) avrà un termine e ne seguirà il rientro in una situazione di normalità, come per il resto d'Italia. C'è piuttosto l'impressione, molto negativa, che l'intero decreto rincorra la confusione esistente e sedimentata, e non affronti con la determinazione che uno Stato consapevole che il suo intervento in sussidiarietà deve dimostrarsi efficace e autorevole dovrebbe invece porre in essere la questione centrale, sinora irrisolta e volentieri innominata, della pesante intromissione della locale malavita organizzata in tutta la filiera della gestione dei rifiuti: questa cancerosa e proterva organizzazione sembra sostituire e lo Stato e le istituzioni locali in un settore, che attiene alla qualità della vita dei cittadini, sia come singoli, sia come collettività. Occorrerebbe tutt'altro spirito a questo testo di legge ed occorrerebbe che il Governo entrasse nel merito di questo specifico tema con una più pregnante azione di positivo condizionamento degli enti locali campani. In carenza di queste condizioni di fondo, questo decreto non sarà certamente l'ultimo ad affrontare tanta problematicità. *(IdV)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, signora Ministro, non appartengo alla schiera di coloro che, per molti versi giustamente, sono ora desiderosi di cavalcare una facile polemica sul mancato avverarsi delle promesse che il Presidente del Consiglio ha fatto - reiteratamente e pubblicamente, dal 2008 fino al mese scorso - in ordine alla imminente e miracolistica risoluzione dei problemi di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania. Non è mio costume utilizzare questi aspetti paradossali e controproducenti della politica degli annunci cui spesso il Governo fa ricorso: voglio invece incentrare il mio intervento su alcune tematiche di fondo, isolando le questioni più delicate e meritevoli di riflessione dalla generalità dei tecnicismi sui quali il Parlamento si è dovuto attardare per anni in virtù di quella che chiamo "statalizzazione" dell'emergenza territoriale, perdendo forse di vista le questioni che la situazione campana può evidenziare a beneficio dì tutto il Paese. Inoltre, sono anche componente della Commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, la quale ha il compito, affidatole dalla legge istitutiva n. 6 del 2009, di svolgere indagini atte a far luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, individuare le connessioni tra queste e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse Regioni del Paese e verso altre Nazioni, i rapporti tra soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo anche in riferimento alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento da parte di enti locali e ai relativi sistemi di affidamento e verificare, infine, la corretta attuazione della normativa vigente, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti pericolosi. Su questo ultimo aspetto, si può affermare che la vicenda ormai quasi ventennale della gestione dei rifiuti nella Regione Campania ha dimostrato senza ombra di dubbio la necessità di una scrupolosa applicazione della legge. Come in altre Regioni, infatti, l'inefficienza del ciclo che si è avuto modo di riscontrare non è quasi mai dipesa da ostacoli di carattere burocratico o amministrativo, quanto piuttosto dalla inidoneità del sistema derogatorio emergenziale a risolvere le problematiche che esso era chiamato ad affrontare in sintonia con gli interessi che la legge tutela: l'ambiente la salute pubblica, l'informazione e la partecipazione dei cittadini, il coinvolgimento delle autonomie territoriali e dei livelli istituzionali interessati. Sono problemi che, certo, continuano ad affliggere la Campania, ma non soltanto essa, come l'attività della Commissione d'inchiesta sui rifiuti ha agevolmente dimostrato. Il regime commissariale, che in un primo periodo ha fatto da tampone all'emergenza, ha contribuito gradualmente, nel corso degli anni, ad alimentarla, sia in Campania che altrove: i meccanismi che esso ha posto in essere hanno deresponsabilizzato gli enti locali e hanno inculcato nella comunità la convinzione che per affrontare un problema gestionale sia necessario disapplicare le leggi, inventare un regime speciale di straordinarietà e con quello gestire procedure di finanziamento e di appalto, affidamento di lavori e nomina delle strutture commissariali, individuazione delle aree da utilizzare, di realizzazione ed esercizio degli impianti. È dunque evidente come ci si trovi di fronte ad un problema di legalità nel senso più stretto dell'espressione, e ciò tanto più nel momento in cui, dopo 16 anni di deroghe alle leggi ambientali ordinarie, ci si trova a riconoscere che è ancora necessario un ulteriore - il sesto - provvedimento di necessità ed urgenza. Paradossalmente, in questo decreto si vuol sancire la fine dell'emergenza, frettolosamente dichiarata a fine 2009 e poi smentita dal permanere di gravi situazioni ambientali in Regione, e contemporaneamente si deroga alla valutazione d'impatto ambientale, al codice dei lavori pubblici e degli appalti e alle norme ordinarie sulla Conferenza di servizi. Dobbiamo allora chiederci: il continuo ricorso a leggi speciali ostacola o favorisce fenomeni di illegalità ed infiltrazione criminale? Contribuisce ad accrescere la fiducia dei cittadini campani nelle istituzioni o mette di fronte le comunità locali a decisioni imposte dall'alto, spesso incomprensibili e comunque mai sufficientemente spiegate a chi vive in quei luoghi? Col mio Gruppo, Italia dei Valori, e il mio partito siamo andati ad incontrare i cittadini a Terzigno e a Chiaiano abbiamo riscontrato un grande problema di fiducia nella politica, signora Ministro e nella pubblica amministrazione. I cittadini hanno bisogno di capire se in quella parte del territorio nazionale, a noi caro, le regole esistono e sono applicate o se, invece, sia destinata a prevalere l'illegalità e, quindi, l'inaffidabilità delle autorità. A fronte di un sistema pubblico commissariale disorganizzato, troviamo un sistema criminale estremamente e capillarmente organizzato. I mezzi di indagine e le strutture investigative devono essere rafforzati. Esistono ordini del giorno in tal senso, anche del nostro Gruppo, di cui auspichiamo l'accoglimento. La sconfitta che lo Stato subisce in una parte del suo territorio, umiliando i suoi cittadini, può trovare risposta solo con una presenza capillare ed efficiente dello Stato su tale territorio, che sia - badate bene - veramente autorevole e non meramente autoritaria. Sono certo importanti gli impianti, ma, se culturalmente non nasce la voglia di capire che la raccolta differenziata, e quindi il ciclo completo del rifiuto, è fondamentale per la crescita sociale, civile ed economica di quel territorio, credo che tutti i nostri discorsi non servano a nulla, o certamente a poco. Ce lo indica la legislazione comunitaria, ce lo impone la normativa nazionale (cito solo il recente decreto legislativo n. 205, che richiede anzitutto la riduzione della produzione di rifiuti), ce lo consigliano le tante esperienze di successo nazionali ed internazionali che hanno sperimentato positivamente tecniche innovative di riciclo totale verso l'obiettivo cosiddetto rifiuti-zero. L'attenzione alla sola impiantistica pesante non ha pagato in tutto il sistema; la disattenzione verso il processo produttivo e verso i materiali *post*-consumo ha invece prodotto pesanti conseguenze. Per questo non voglio neanche entrare nel merito dei temi di Acerra e di Salerno e dei necessari controlli che occorre porre in essere per evitare che la criminalità, oltre alle discariche abusive, si occupi anche dei lavori per la realizzazione dei cosiddetti termovalorizzatori. So solo che un vero piano dei rifiuti, un vero decollo della legalità è l'unica speranza per non avere, da qui alla fine della legislatura, altri sei o sette decreti-legge. Legalità significa anche rispettare, come l'Unione europea ci chiede, i parametri di tutela della salute dei cittadini, di qualità dell'aria, delle falde acquifere, dei suoli; il che significa, per esempio, non bruciare nei termovalorizzatori i rifiuti organici, che devono essere smaltiti con altre tecnologie che ancora ci rifiutiamo di utilizzare. C'è poi il problema della tracciabilità dei rifiuti, e quindi del sistema di monitoraggio SISTRI, a lungo rinviato, e della sua versione campana (SITRA). Di questi aspetti il decreto non si occupa, e perciò si conferma carente e debole. La politica e le istituzioni devono offrire servizi efficienti alla cittadinanza, essere totalmente impermeabili all'illegalità e alla presenza malavitosa, evitare assolutamente che su temi tanto delicati ci si divida lungo linee non trasparenti, secondo interessi occulti che si confrontano sopra il ruolo politico e amministrativo sul territorio. Credo, infine, che il vero problema che il vero problema sia capire chi ostacola il decollo economico e civile di quella realtà. Rispondendo a quella domanda si troverà anche la risposta alle ragioni dei ritardi, spesso incomprensibili, che l'organizzazione della raccolta differenziata e del ciclo dei rifiuti hanno incontrato in particolare, ma non esclusivamente, in questa Regione.

a quando la fine dell'emergenza? Il decreto sembra segnare la fine di un'emergenza. Il Presidente del Consiglio continua a dirci che è tutto risolto, va tutto bene, ma questo decreto conferma ancora una volta che

ma è davvero finita questa emergenza? Davvero va tutto bene, come si ostina a dire il Presidente del Consiglio? Io credo di no. Un conto sono allora gli annunci televisivi, un conto poi gli atti conseguenti, anche se questo atto, per l'ennesima volta, risulta a mio parere inadeguato e per certi aspetti confuso. La seconda questione che vorrei affrontare riguarda il tema della sicurezza e autorevolezza del sistema. In questo decreto si fanno sparire alcune localizzazioni di discariche. Non voglio entrare nel merito, può essere anche giusto, ma non è che ogni vota possiamo fare un elenco di discariche, poi l'elenco cambia e se ne introduce una nuova. Se fossi un cittadino della Campania mi chiederei: con quale criterio viene scelta una localizzazione nel mio Comune? Posso fidarmi di un sistema che continuamente cambia gli elenchi? Allora, la questione dell'autorevolezza nella scelta dei siti degli impianti è fondamentale. Poi ci lamentiamo che i cittadini, e magari i sindaci, scendono in piazza contro una localizzazione. Ma se le localizzazioni cambiano continuamente che fiducia può esserci Entrerò poi nel merito di una questione tecnica che dimostra come questo sia davvero un problema consistente. perché cambiare continuamente localizzazione? Perché continuare a redigere elenchi che poi mutano di volta in volta? Ebbene, gli elenchi mutano perché alcuni cittadini sono più furbi di altri e la loro protesta è più ascoltata di quella

i cittadini che abitano in quel territorio. Questo è un problema che va risolto. Tutto il Sud (mi si permetta), non solo la Campania, ha questo problema: enti locali che si ribellano a un sistema di gestione dei rifiuti che ogni volta viene

Non volete credere a questa minoranza brutta, sporca e cattiva. Bene, credete almeno alla relazione tecnica redatta dagli Uffici del Senato,

dopo il declassamento a "frazione umida" (CER 19.05.01) (...) a causa della scadente qualità del materiale in uscita dagli impianti stessi al fine di destinarlo a copertura delle discariche» e a bonifica delle cave, discariche e quanto altro, È vero che è stata fatta una sperimentazione su questo tipo di rifiuto, però il decreto non dà alcuna garanzia che il cambio del codice dei rifiuti avvenga dopo che tutti i rifiuti siano stati sottoposti alla procedura di biostabilizzazione.

rifiuti nelle discariche, dentro le cave, eccetera. Non si possono fare operazioni come queste. Torno a ripetere, è la relazione tecnica degli Uffici del Senato...

intervengo per esprimere il mio apprezzamento per questo intervento del Governo,

la data di nascita dell'atto di commissariamento è l'11 febbraio 1994, come è stato ricordato

che ponesse come precondizione un richiamo alla solidarietà istituzionale e a tutte le istituzioni affinché ciascuna facesse la propria parte. Io mi sono veramente

la prova è che i rifiuti sono in mezzo alla strada? Oppure, che senso ha dire che in alcune zone di un certo rione si fa la raccolta per bene a differenza di altri rioni, per giustificare magari alcune inadempienze? Bisogna dire la verità: se un'amministrazione non fa il suo dovere, bisogna dirlo, perché è un problema che poi scoppia e che ci troviamo a gestire con tutte le emergenze

che a Napoli la gestione dei rifiuti non funziona perché c'è la malavita organizzata. Certo, ci sono state delle indagini giudiziarie che sono terminate con arresti, però

Per esempio, i due termovalorizzatori di Salerno e di Napoli dove sono? Perché non ci sono ancora? Chi li deve Voglio richiamare e ringraziare il presidente della Provincia di Salerno. Dopo anni di immobilismo, di palleggiamento di responsabilità, il termovalorizzatore sarà realizzato purché il Comune di Salerno riceva 30 milioni di euro.

che se non ci sono gli impianti, il problema non si risolverà. Allora sarà il presidente Berlusconi o un altro Presidente del Consiglio che dovrà intervenire, sarà la Protezione civile, il Ministero dell'ambiente, ma questi rifiuti che vengono prodotti dai cittadini campani chi li deve smaltire?

si sintonizzavano con la legge regionale, ed è giusto. Se la Regione ha un governo regionale, se quel governo regionale si è dato una legge per per regolamentarsi, per gestire questo problema, è giusto che ci sia una sorta di rapporto con quella legge. con quella legge. Il presidente Caldoro, il nuovo governo regionale questo deve fare: deve studiare, deve mettere in campo una capacità elaborativa, un nuovo piano per la gestione dei rifiuti.

Allora, per sgombrare il campo dagli inutili e spesso dannosi tatticismi, preannuncio fin d'ora il voto favorevole sul provvedimento in esame. Non certamente come voto di fiducia all'operato del Governo, ma solo e soltanto come voto di speranza per i campani, e i napoletani in particolare.

Fu anche grazie a questo che nella mia Regione il dato elettorale fu quanto mai soddisfacente per le vostre liste ma oggi, se la situazione non fosse tragica, ci sarebbe solo da sorridere. Oltre al danno continuato, ci fu pure la beffa perché allora, come oggi, l'Unione europea, per tramite dei suoi ispettori, ci ha notificato che il problema non è stato risolto; anzi, ci hanno detto che dopo due anni la situazione non è molto diversa. I rifiuti sono ancora per strada, non c'è una rete integrata per la gestione della raccolta differenziata, non c'è un ciclo virtuoso. Insomma, non c'è niente, se non l'immondizia per le strade. Allora, nel ricordare a me stesso un motto che mi è caro, che risale alle mie esperienze giovanili e che testualmente recita: «Non chiedo il dove, non chiedo il quando e non chiedo il perché», apostrofai la vostra inerzia nel non voler il dove, il quando e il perché si sarebbero smaltite le migliaia di tonnellate di rifiuti per strada e, fatto ancor più grave, le milioni di ecoballe che non si sa quando e dove si dovranno smaltire. Ancora oggi, a distanza di due anni e mezzo, sono ancora qui a chiedervelo, nella speranza che il Governo ci sappia dare un'indicazione, sia pure di massima. Dove le metterete, tenuto conto che

Potremmo anche darvi qualche consiglio, ipotizzando ad esempio la sostituzione del combustibile fossile con il combustibile rinnovabile proveniente dai nostri rifiuti, il cosiddetto CDR. In Italia si producono 35 milioni di tonnellate di rifiuti. Di questi, meno della metà vengono raccolti separatamente e bruciati nei forni inceneritori. Rimangono, quindi, circa 20 milioni di tonnellate di rifiuti indifferenziati.

Ci avete mortificato ricordandoci a ogni piè sospinto che detenevamo il controllo della Regione, quella Regione allora governata dal centrosinistra e da Antonio Bassolino,

dimenticando volutamente che la questione dei rifiuti è ormai un fatto che attiene alle Province, le stesse da voi amministrate. Oggi siamo qui a chiederci chi è che farà uguale atto di coraggio oppure se dovremo continuare a d aspettare le discese in campo di Berlusconi che, con cadenza quasi settimanale, ha inondato i giornali di spot pubblicitari sulla risoluzione del problema, risultato poi assimilabile soltanto a una bufala, argomento di cui in Campania siamo esperti. Oggi, dopo quasi due anni, le cose sono cambiate. Molte Province sono nelle vostre mani. La Campania, seconda Regione per numero di abitanti, è nelle vostre mani. Nonostante ciò, si assiste al teatrino dei rimbalzi di responsabilità, alla guerra di potere e alla voglia tutta personale di fare affari con l'immondizia.

ma se questo provvedimento serve a riaccendere la speranza, al di là delle posizioni politiche e delle critiche alla maggioranza, non possiamo non far prevalere, per il ragionevole dubbio che almeno qualcuna di queste disposizioni possa favorire o almeno alleggerire il peso che questa tragicommedia ha sulle sorti di Napoli - che poi viene strumentalizzata a livello nazionale ed anche all'estero

finalmente riusciamo ad addentrarci nei meandri dei rifiuti di Napoli. Spero che poi affronteremo anche la questione nazionale, perché non possiamo parlare di Napoli se non parliamo anche della questione nazionale dei rifiuti, per motivi che adesso mi accingerò ad

Quando si parla di ciclo integrato dei rifiuti, si intende il sistema volto a gestire l'intero processo dei rifiuti, dalla produzione alla sorte finale, e comprende la raccolta, il trasporto, il trattamento e, quindi, il riciclaggio e lo smaltimento attraverso una rete integrata di impianti. Il sistema di gestione dei rifiuti è individuato da diversi processi e dalle loro interrelazioni che riguardano la raccolta, la separazione, il trattamento e lo smaltimento finale. I processi di impianti e le attività sono operazioni associate alla gestione dei rifiuti. Sul quadro europeo la gestione dei rifiuti in Italia fa riferimento ai programmi della Comunità europea, mentre nella legislazione dei Paesi membri risulta prioritaria l'azione della minimizzazione dei rifiuti secondo varie gerarchie dei lavori che prevedono sia la prevenzione che poi lo stesso riciclo. La definizione di minimizzazione dei rifiuti, intesa come riduzione della loro quantità e nocività per l'ambiente, comprende sia la prevenzione, sia la riduzione alla fonte, sia il riutilizzo del prodotto e lo stesso riciclaggio. I principi riguardano la gerarchia degli interventi - il principio dell'autosufficienza e della prossimità in materia di smaltimento - e riguardano, sempre a livello europeo, la regola del chi inquina paga (dopo

Fatto sta che l'Europa, o meglio molti Paesi d'Europa, hanno raggiunto un livello ottimale; in Italia la situazione rispetto a questi virtuosismi europei è, più o meno, secondo i dati delle riviste specializzate, al 50 la metà dei nostri rifiuti finisce in discarica. Il problema certamente non è affrontato dal decreto-legge n. 196 del 2010, 2010, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della Regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Le amministrazioni territoriali devono farsi carico e assumersi le proprie responsabilità, ma non è stata un'invenzione di questo Governo. Lo stesso sindaco di Napoli, in un'intervista a «la Repubblica» del 19 ottobre 2010, invocava questo tipo d'intervento. Il sindaco di Napoli non è Napoli non è di centrodestra, così come non è stato di centrodestra il governo della Regione Campania. Se andiamo a vedere tutto ciò che è successo, ci rendiamo anche conto che da 20 anni si parla di rifiuti in Campania. Questi 20 anni sono trascorsi inutilmente, perché il problema non lo abbiamo risolto. Oltre a non risolvere il problema, molte volte attribuiamo delle responsabilità alle cosiddette ecomafie che, secondo un revanscismo che riguarda che riguarda un fatto secessionistico, interessano soltanto la questione meridionale. Se però andiamo a fare uno *screening* di quanto successo in questi anni, certamente non possiamo attribuire responsabilità ai campani perché le loro discariche sono ormai

quali sono gli scandali nazionali che molte volte qualcuno vuole attribuire alla Campania o allo stesso meridione in nome delle questioni dell'ecomafia. È troppo facile nascondersi dietro la malavita locale quando sappiamo molto bene

denominato Fenice, che cogenera contestualmente 38.000 megawatt di energia elettrica.

potremmo quasi esaurire l'intero ciclo dei rifiuti depositati in ecoballe in qualche luogo a Napoli, senza dire quali sono poi le conseguenze. È troppo

oggi ci troviamo di nuovo nelle stesse condizioni. Dopo 16 anni di emergenza, a circa un anno dalla propagandistica proclamazione della fine dell'emergenza, ci si sarebbe attesi una legge ordinaria e organica, capace di gettare le basi normative per avviare finalmente una politica strutturale corretta ed efficiente di gestione a lungo termine di quei materiali che potrebbero costituire preziose risorse, ma di cui ci si preoccupa assiduamente solo quando - come ho detto - emergono problemi in merito al loro smaltimento come rifiuti. Abbiamo, invece, l'ennesimo decreto-legge che non si discosta minimamente dal solco avviato negli anni più o meno recenti, che si è dimostrato inconcludente e antieconomico, peggiorando sensibilmente la situazione proprio negli anni più recenti. È la sola constatazione della pochezza dei risultati, a fronte della enormità delle risorse spese, avrebbe dovuto indurre il Governo a cambiare radicalmente registro, ribaltando l'approccio seguito finora. Continua a mancare una visione complessiva del ciclo completo dei rifiuti, basandosi tutti i piani e i provvedimenti che ci vengono proposti esclusivamente sulla fase finale della vita dei prodotti e, quindi, sull'impiantistica pesante (discariche e impianti di combustione). La mancanza di investimenti e di idee su tutta la prima parte non solo ci costringe mediamente ogni sei mesi a tornare sull'argomento senza mai risolverlo, ma è retaggio di una impostazione ormai vecchia che l'Europa ha già abbandonato da tempo. Su questo punto abbiamo presentato l'ordine del giorno G102, che impegna il Governo a tener conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti e a non trascurare gli aspetti del compostaggio e del riciclo in un quadro finalizzato all'abbattimento della quantità e pericolosità dei materiali già prima della fase del consumo. Lo stesso ordinamento italiano si è recentemente dotato di un decreto legislativo che recepisce la direttiva 2008/98/CE in cui la gerarchia delle azioni e delle misure appare praticamente capovolta rispetto a quella che il decreto in esame, al pari di quelli che lo hanno preceduto, stancamente porta avanti. L'obiettivo «rifiuti zero» non appare neppure tra le righe del testo; la raccolta differenziata domiciliare è ancora trattata come una sorta di Cenerentola, lasciata priva di adeguati investimenti e di più forti misure sanzionatorie per i Comuni inadempienti. Piuttosto, nel recente passato, si è pensato bene di sanzionare i Comuni virtuosi che esistono anche in Campania e sono più numerosi di quello che spesso si immagina. Si è infatti confermata, salva una proroga introdotta alla Camera con emendamento dell'opposizione, la tesi di fondo secondo cui la provincializzazione delle competenze sul ciclo dei rifiuti costituisce un'ottima soluzione all'emergenza. In tal modo, si sottrarranno risorse e funzioni anche a quei Comuni, come ho detto, che hanno raggiunto e ampiamente superato gli obiettivi di raccolta differenziata per affidarli ad enti e società che mai si sono occupati di questa materia. Tutto ciò non è politicamente criticabile: è irragionevole, è privo di senso. Eppure si persevera nell'errore, salvo concedere una proroga al regime attuale che evidenzia la piena coscienza dell'errata impostazione legislativa. Si è detto della provincializzazione: non è questa la sede per rievocare i contrasti all'interno della maggioranza che questo decreto ha comportato, culminati, dopo un contrasto fortissimo un contrasto fortissimo tra Presidenza della Regione e Presidenze provinciali, nelle annunciate e poi ritirate dimissioni del Ministro delle pari opportunità. Tensioni mai sopite, se è vero che proprio su una questione connessa alla tracciabilità dei rifiuti nell'ambito di un altro provvedimento il Ministro dell'ambiente ha trovato le ragioni per lasciare il partito del Presidente del Consiglio. La tracciabilità è una delle altre grandi assenze del decreto: i sistemi di monitoraggio della origine e della destinazione dei rifiuti si susseguono uno dopo l'altro, ed anzi si duplicano e si sovrappongono. A livello nazionale c'è il SISTRI, e mi dispiace che non sia presente il Ministro, perché a livello campano esiste il SITRA, che riguarda anche i rifiuti urbani. Il SISTRI è stato più volte rinviato, da ultimo il 28 dicembre scorso, per veri o presunti problemi di applicabilità tecnica. Del SITRA non si riesce ad avere una messa a regime piena e completa. Nel frattempo, sia per l'uno che per l'altro sistema sono state spese ingenti risorse e non è pertanto sostenibile continuare in tale indecisione senza nascondersi i problemi che si possono determinare sul controllo e la prevenzione delle illegalità nei traffici di rifiuti.

Allo stesso modo, invitiamo il Governo a rafforzare gli strumenti di indagine e contrasto alla criminalità, tenendo conto del fatto, come ricorda l'ordine del giorno G103, che la direttiva 2008/99/CE impegna anche il nostro Paese a rafforzare la tutela penale dell'ambiente. Né si parla, nel decreto, delle famose ecoballe, quegli agglomerati che di ecologico non hanno nulla, ma che ammontano a molti milioni di tonnellate di peso, occupano vasti spazi e non possono essere trattate termicamente perché ottenute in modo non conforme alla normativa nazionale e comunitaria vigente. Su questo punto, e sulle conseguenti attività di ripristino e bonifica, abbiamo presentato un altro ordine del giorno. Ma se sono numerose le assenze, quelle che potremmo definire le norme fantasma in questo decreto, ciò deriva forse dal fatto che il provvedimento stesso per molti giorni è stato un decreto fantasma. Il 18 novembre 2010 il Consiglio dei ministri approvava con la irrituale formula "salvo intese", quindi con un testo non definitivo e suscettibile di ulteriori modifiche, il decreto-legge in esame. Il nodo principale, a conferma del capovolgimento delle priorità rispetto alla normativa comunitaria, era legato ai termovalorizzatori, e soprattutto alle procedure con cui affidare la gestione della loro costruzione. Su questa lite intorno ai poteri del Presidente della Regione, è nata la crisi, tutta interna, del PdL. Su questo punto sappiamo, dagli organi di stampa, che si è arrivati ad una seconda stesura del decreto. Intanto, dopo alcuni giorni, la Presidenza della Repubblica informava con un secco comunicato stampa che «il Presidente non ha ricevuto e non ha potuto quindi esaminare il testo del decreto-legge sulla raccolta dei rifiuti e la realizzazione dei termovalorizzatori». Solo dopo un ulteriore sollecito il Presidente ha potuto visionare il testo sul quale, come è noto, ha avanzato anche rilievi tecnico-giuridici afferenti proprio il rapporto Provincia - Regione. Tra l'uscita da Palazzo Chigi e l'arrivo al Quirinale, dunque, sono passati dei giorni in cui il testo fantasma cambiava forma e contenuto.

settori importanti nel Sud che ci consentono di portare sviluppo economico ed occupazionale: il turismo e l'agricoltura. Li stiamo distruggendo. Stiamo distruggendo l'occupazione nel Sud e tante famiglie e tanti giovani che sperano che un Parlamento governi, e bene, per farli rinascere.

da far male un paio di anni fa, si è riproposta in modo da fare ancora male la vigilia di Natale. In questi 15 lunghi anni si sono succeduti si sono succeduti Governi nazionali e locali, non sono servite decretazioni d'urgenza, non è servita la Protezione civile, non l'Esercito, non le deroghe alle disposizioni in materia ambientale e igienico-sanitaria, non le deroghe alla prevenzione incendi, alla sicurezza sul lavoro, urbanistica, financo ai beni culturali ed al paesaggio; perfino la disciplina dei termovalorizzatori è stata modificata per porre fine a questa tragedia. Sono state introdotte forme di vigilanza nei confronti degli enti locali. È stata prevista una disciplina sanzionatoria più incisiva per i Comuni inadempienti. Tutto questo non è bastato e non è servito a liberare Napoli e la sua Provincia da un'emergenza che ne offende la dignità individuale e collettiva.

non si vota neanche quello che in questo momento sembra servire di più, come altri hanno fatto, appartenendo a quei Gruppi che sostanzialmente cercano di valutare passo per passo le iniziative che possono essere utili al Paese, ci accingiamo a votare positivamente questo decreto.

per lo smaltimento dei rifiuti, ma credo debba riguardare ciascuno di noi, per cercare di capire se ciascuno di noi può, nel contesto in cui si trova e in cui esercita una sua funzione, essere solidale con un dato che, a mio avviso, non è soltanto campano. Assistono ai nostri lavori studenti di quelle aree, studenti campani, che sono prima di tutto cittadini di questo Paese: questo è un problema che mi riguarda come cittadino di questo Paese,

Mi sono ritrovato in parole dette precedentemente, che certo non negano la realtà di una criminalità organizzata che su questo marcia straordinariamente bene: ma le responsabilità non possono essere pensate e declinate soltanto al meridionale. Certo è che se quel che percepito è, la sfiducia è molto forte, ed è in essa che sostanzialmente si trova il tessuto fertile, l'*humus* straordinariamente valido per l'inserimento dell'attività illegale.

Orsi. Credo perciò che abbiamo davvero una gran bella responsabilità. Sarà forse proprio perché, scoutisticamente parlando, sono stato abituato a lasciare pulito il prato in cui bivaccavamo, dovremmo immaginare così questo nostro passaggio: lasciare pulito il tempo che noi viviamo, per non lasciare sporcizia ai ragazzi che ci seguiranno e per non concludere tutto con un «io speriamo che me la cavo».

è stato desolante quello che è successo quest'anno, tanto più che era ampiamente prevedibile. Il 22 settembre dell'anno passato abbiamo presentato un'interrogazione, nella quale si annunciava che l'emergenza rifiuti in Campania, particolarmente a Napoli, continuava. Le cause di questa continua emergenza sono varie; prima di tutto vi è la cessazione del commissariamento. È, infatti, chiaro che il commissariamento è stato un modo per evitare - almeno

società degli imprenditori Gavioli, ENEL Ambiente, che effettua la raccolta della spazzatura in due terzi della città di Napoli, raccogliendo quindi 1.000 tonnellate al giorno, al giorno, e che minaccia la sospensione del servizio in quanto vanta un credito di 13 milioni di euro dalla società «Asia» del Comune

una notte, si sono ammalati 68 conduttori di camion della raccolta della spazzatura, tutti presi da un'epidemia fulminea. Poi i camion che questi signori guidavano sono rimasti fermi

tonnellate al giorno, si è accumulata per tre-quattro giorni, con il risultato che la città è stata ricoperta di rifiuti. In tale situazione si sono naturalmente inseriti tutti i vari interessi della camorra e dei locali, che hanno inscenato le solite manifestazioni. Quindi, la crisi di Napoli si è allargata alla crisi delle discariche,

Questa situazione, malgrado il finanziamento di 7 milioni di euro erogato dai fondi del Programma operativo regionale (POR), non è avviata a soluzione, anzi, gli impianti previsti nell'area del centro di compostaggio di via

Presidente, componenti del Governo, colleghi, è certo difficile per un esponente della Lega Nord parlare dei problemi della città di Napoli: sarebbe come sparare sulla Croce Rossa. Sono sicuro che alcuni di voi si aspettano dichiarazioni magari folli, ma vi dico subito che non sarà così. Curioso, vero? A cosa servirebbe parlare di commissari e altro, come ho sentito alcuni colleghi fare, oppure riprendere quei colleghi che hanno voluto affermare ancora una volta che il disastro di Napoli è colpa

sono avventurieri che abitano al Nord e che approfittano di tali situazioni, di certo non ne possiamo essere noi i responsabili. Dunque, come dicevo, voglio esporre un vero ragionamento, che mi ha sempre confortato e supportato da quando sono entrato in Parlamento nell'ormai lontano 1987. Non ho mai pensato e vissuto da individualista. Sono convinto che un uomo non può realizzarsi integralmente senza volersi impegnare nella realtà sociale, così difficile da realizzare nella nostra società. La cultura federalista, che da sempre ho approfondito e studiato, mi ha fatto capire che l'uomo si può definire federalista quando si sente libero e impegnato, ma anche autonomo e solidale. Deve così vivere una tensione di amore fra questi due poli, il privato e il collettivo, tra queste due responsabilità, la sua vocazione e il Paese in cui vive, infine, tra questi due amori, quello che deve a se stesso (e dunque alla sua famiglia, alla sua comunità e alla sua città) e quello che deve al suo Paese È un uomo chiamato a vivere una continua tensione d'amore tra un ambito di dibattito creativo e un ambito di dialogo

bastato uscire dalla stazione ferroviaria per rendermi conto del grande disastro. Ho fatto un giro anche nella città e lo spettacolo era simile in tutti i quartieri. Quelle immagini hanno evocato in me le foto dell'ultimo conflitto mondiale, dove i bombardamenti arrecarono crolli e le macerie risultavano sparse lungo le strade e le piazze. Ho colto questa similitudine. Ora, come allora, Napoli ha bisogno di cittadini responsabili, di persone ricche di spirito federalista che amino la loro città, la propria persona. Solo così questa bella città potrà rinascere. La ricetta è investire nelle persone. Non saranno né le giunte di destra, né di sinistra, né i decreti, né i commissariamenti che risolveranno i problemi, ma la coscienza dei napoletani, di tutti i napoletani. Bisogna far capire loro che ci sono altre ricette come, per esempio, la ricetta dell'amore per le proprie cose e per la propria città. Nel Paese è il pensiero e l'organizzazione federalista che renderà tutti tutti più responsabili, ma anche più liberi. È sulla bocca di tutti che il male di questa città è la camorra,

Lavoriamo per dare ai cittadini di Napoli la speranza di poter vivere in libertà e di poter rimettere a posto la loro città.

dei rifiuti in Campania con un spirito non strumentale, non pregiudiziale ma con una voglia di trasparenza, di realtà e di verità credo debba sicuramente informare i nostri lavori. Ed è proprio perché vogliamo seguire questo percorso e accettare questo appello ad essere seri e responsabili che credo che alcuni aspetti di questo decreto debbano essere sottolineati criticamente. Se pensiamo che - come è stato detto da da tanti oggi in quest'Aula - non ci sia una sola responsabilità, dalla parte del centrosinistra, e invece capacità miracolistiche da parte dell'attuale Governo,

all'ente locale di turno le responsabilità della crisi, compresa la crisi di questi giorni, che non è apocalittica come l'ha raccontata

trasferiva la competenza dell'ordinario agli enti locali. Troppo precipitosamente e con pasticci su pasticci è stata dichiarata la fine dell'emergenza e il ritorno all'ordinarietà, che non è mai cominciata perché non c'è mai stato un percorso di razionalizzazione delle competenze e delle funzioni delle amministrazioni locali, che sono state chiamate a subentrare ai commissari senza essere dotate di strumenti, risorse e di una legislazione adeguata. L'unica condizione subentrata all'emergenza è l'emergenza che è ancora sotto gli occhi di tutti noi. È una situazione complessa quella della gestione dei rifiuti.

mi permetterò di sottolineare alcuni ulteriori aspetti nell'illustrazione dell'ordine del giorno e degli emendamenti che abbiamo presentato al decreto.

senatori, il decreto-legge n. 196 del 2010, così come emendato e modificato dalla Camera dei deputati, viene sottoposto alla nostra approvazione per la definitiva conversione in legge. Lo stesso rappresenta per la Regione Campania l'ulteriore e speriamo ultimo intervento normativo all'indomani della cessazione dello stato di emergenza ed è nato dalla necessità di integrare e, laddove necessario, modificare quanto previsto dalla legge n. 26 del 2010 (legge di conversione del decreto-legge n. 195 del 2009). La citata legge n. 26 del 2010, nella fase immediatamente successiva alla cessazione dello stato di emergenza, ha disciplinato e favorito il passaggio dalla fase emergenziale a quella ordinaria del ciclo integrato dei rifiuti nella Regione Campania, articolando un insieme di norme che, come genesi, trova fondamento nella legislazione regionale, con particolare riferimento alla legge n. 4 del 2007, che ha individuato nell'ente Provincia l'ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti. Tuttavia, nella prima applicazione della legge, che pure tanto ha contribuito al rientro in regime ordinario delle attività, è stata evidenziata la necessità di meglio chiarire e stabilire in modo inequivocabile i percorsi amministrativi attraverso i quali procedere ad una corretta gestione dell'intero sistema. Questo, per due ordini di motivi. Il primo, per le problematiche che si riscontrano nelle varie Province, e parlo anche nella veste di presidente della Provincia di Avellino. A questo proposito apro una parentesi sulla cosiddetta emergenza: per il ciclo rifiuti, è assolutamente autonoma e virtuosa; raggiunge una quota di raccolta differenziata di circa il 60 per cento e ha concesso e continua a concedere una quota di solidarietà a Napoli e alla sua Provincia, dove purtroppo non si raggiungono quote di raccolta differenziata significative, trasferendo così il problema sulle altre Province della Regione. Dicevo che le problematiche sono di natura diversa, atteso che le stesse derivano essenzialmente da quanto ereditato dalle precedenti gestioni, e spesso contrastanti. In secondo luogo perché, trascorso un anno dalla cessazione dello stato di emergenza, le necessità dei vari enti derivano dal modello organizzativo prescelto e differiscono in virtù di quanto allo stato hanno realizzato e di quanto nel breve dovranno realizzare. Quindi, è necessario procedere ad un'attenta analisi dell'intero impianto normativo, evidenziando nello specifico le norme che attualmente risultano carenti e quindi necessitano di interventi migliorativi e ciò che va regolamentato ulteriormente per consentire all'intero sistema, enti locali compresi, di dotarsi degli strumenti opportuni per far sì che il sistema decolli e vada a regime. In prima istanza è necessario affermare senza possibilità di smentite che il sistema impiantistico della Regione Campania è inadeguato, per diversi ordini di motivi: motivi: per la mancanza di siti di discarica essenziali ad un efficiente sistema; per la mancanza di siti di compostaggio idonei a ricevere un aumento della raccolta di organico, che in alcune Province ha raggiunto livelli soddisfacenti; per l'impiantistica di supporto alle raccolte: impianti, termovalorizzatori e/o inceneritori a valle del sistema, che ad oggi risultano insufficienti. Ma per l'individuazione dei siti dove collocare questi impianti, per la progettazione e costruzione degli stessi è necessario che vengano conferiti a diversi soggetti, tra cui i presidenti delle Province, straordinari, così come già previsto dall'articolo 11 della legge n. 26 del 2010 sino al 30 settembre 2010. Di qui la necessità di prorogare i poteri straordinari ai presidenti delle Province per la parte di competenza delle amministrazioni provinciali sino al 31 dicembre Sarebbe, quindi, opportuno prorogare almeno di un ulteriore anno i poteri in capo al presidente della Provincia, così come già normato dall'articolo 11 della legge n. 26 del 2010. Anche i servizi di raccolta gestiti dalle società provinciali richiedono una regolamentazione tecnico-amministrativa che dal punto di vista economico dia certezza di funzionalità. Le norme attuali non consentono di garantire i flussi finanziari alle società provinciali, le quali lamentano di non avere nella loro disponibilità la certezza dell'incasso delle prestazioni. L'attuale sistema del recupero dei costi attraverso la TARSU non appare lo strumento idoneo a far sì che il soggetto gestore abbia la certezza dell'incasso, dovendosi accollare eventuali morosità e la tempestività degli stessi, atteso lo sfasamento temporale tra incassi e pagamenti. A ciò potrebbe porsi rimedio considerando che le prestazioni delle società provinciali sono rese a favore dei Comuni, i quali devono provvedere al pagamento di quanto dovuto a prescindere dall'avvenuto incasso dei ruoli TARSU. Nella sostanza, il Comune si deve rendere garante e parte attiva nel procedimento amministrativo che regola il rapporto finanziario tra committente e prestatore di servizi. Un discorso diverso andrà disciplinato in presenza del sistema tariffario qualora se ne renderà possibile l'applicazione. Sempre in tale ottica è il caso di sollecitare i Comuni affinché l'emissione dei ruoli, annualmente, avvenga non oltre giugno. Ciò garantirebbe maggiore liquidità agli stessi Comuni per adempiere alle obbligazioni assunte nella gestione del servizio. Va inoltre affrontata la problematica, più volte evidenziata, della necessità per le Province che ne hanno l'opportunità, di consentire il finanziamento delle attività del ciclo dei rifiuti con l'avanzo di amministrazione. è la problematica riguardante la fase liquidatoria dei consorzi di bacino *ex* legge regionale n. 10 del 1993, rispetto alla quale è necessario disciplinare dettagliatamente il percorso amministrativo-contabile per addivenire alla definizione dei piani di liquidazione. Sarebbe auspicabile l'inserimento di norme che prevedano il blocco degli atti giudiziari in corso, che individuino le fonti di approvvigionamento per la definizione dei piani di liquidazione, che individuino il percorso amministrativo-contabile da seguire nel procedimento di accertamento delle masse creditorie e debitorie, nonché nella redazione del piano di liquidazione. Per concludere, e con un occhio al passato, è necessario un intervento risolutivo sulle problematiche economiche che riguardano l'incapacità dei Comuni a fare fronte alle debitorie pregresse. A mio parere è necessario un intervento del Ministero dell'economia e delle finanze che sostenga gli enti locali nell'adempimento delle obbligazioni, sorte nel periodo emergenziale. Non credo - e concludo davvero - che oggi i Comuni non siano in grado di sostenere il costo dell'attuale servizio, ma è certo che quegli enti che nel corso degli anni precedenti si sono avvalsi della facoltà, agli stessi concessa per brutale permissivismo, di non corrispondere quanto dovuto, oggi si trovano nella condizione di non poter adempiere alle proprie obbligazioni passate e a quelle della gestione corrente, con conseguenze facilmente immaginabili.

Presidente, ringrazio i colleghi per gli interventi svolti, che, al di là delle posizioni politiche,

apre una nuova finestra"). Onorevoli colleghi, comunico che, previ accordi intercorsi tra i Gruppi, l'ordine del giorno dell'odierna seduta pomeridiana è integrato con la votazione per l'elezione di nove componenti effettivi e nove componenti supplenti della delegazione presso le Assemblee parlamentari del Consiglio d'Europa e dell'Unione dell'Europa occidentale I Gruppi saranno previamente informati dell'orario in cui si procederà al voto, che avrà luogo a scrutinio segreto con procedimento elettronico su lista bloccata.

colleghi, ieri sera «Striscia la notizia» ha mandato in onda in un servizio le proteste di alcuni risparmiatori del Banco emiliano romagnolo il piccolo istituto bolognese in amministrazione straordinaria che lo scorso 6 dicembre ha congelato i depositi, negando ai clienti la possibilità di ritirare dai propri conti soldi, titoli ed altri strumenti finanziari, già oggetto dell'atto di sindacato I commissari straordinari del Banco emiliano romagnolo, previa autorizzazione della Banca d'Italia, hanno deliberato la sospensione del pagamento delle passività di qualsiasi genere e della restituzione degli strumenti finanziari alla clientela, ai sensi dell'articolo

il Governatore della Banca d'Italia Draghi ha nominato commissario della banca il signor Fernando De Flaviis, con gravissimi problemi giudiziari (oggetto degli atti di sindacato ispettivo 4-01956 e 4-03889),

"Notizie di reato modello 21", relativamente al periodo in cui ricopriva la carica di direttore generale della Cassa di risparmio della Provincia di Teramo, banca Tercas, tra il 1998 ed il 2005; Non conosco le ragioni della mancata revoca del commissario De Flaviis da parte del governatore Draghi e se ciò non sia stata la principale causa del congelamento dei depositi a distanza di 16 mesi dalla data del commissariamento, né posso pensare che tra i criteri di onorabilità per gestire le banche in crisi la Banca d'Italia acquisisca

la prova provata di uno scandalo insopportabile da parte del governatore Draghi e di una Banca d'Italia che continua a non rispondere ad alcuno del suo operato, favorevole agli esclusivi interessi dei banchieri e proprio per questo contro i diritti e gli interessi dei risparmiatori. Il Governo non può continuare a fare finta di niente, ha l'obbligo di pretendere dal signor Draghi di conoscere quale fine abbiano fatto i risparmi dei clienti della BER e perché abbia nominato commissario un signore indagato per il reato di usura, anche se ciò

Si tratta di una richiesta di informazioni, ma anche di un sollecito allo stesso Ministro ad inviare degli ispettori presso il Comune di Salerno in cui sono stati denunciati una serie di falsi in bilancio sui quali bisognerebbe